Comunico, come già indicato per le vie brevi ai Gruppi, che la seduta sarà sospesa fino alle ore 12,15 per consentire la presentazione, entro le ore 12, di eventuali subemendamenti agli ulteriori emendamenti del Governo trasmessi nella serata di venerdì 22 febbraio. La seduta è sospesa.

anche ai nostri uffici, per elaborare in maniera appropriata la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del Governo e della maggioranza. Quanto però intendo chiederle, signor Presidente, è che i lavori dell'Assemblea non vadano avanti

Lei lo sa bene, Presidente, perché il suo intervento ha solo parzialmente emendato la continua rottura del dibattito democratico che sta avvenendo all'interno dell'Aula e delle Commissioni.

e voi ascoltare per risparmiare tempo, perché questo è avvenuto fino adesso. È avvenuto per la legge di bilancio e per la riduzione del numero dei parlamentari. Abbiamo una maggioranza così silenziosa da essere muta per non perdere perdere quel tempo che - colleghi - si chiama democrazia e rappresentanza popolare. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Vi do una notizia, colleghi, e in questo provvedimento in particolare questa notizia è importante: il popolo non lo rappresentate solo voi, ma esiste una porzione

vorremmo anche che voi ci rispondeste, come finora non è stato fatto. E vorremmo, se possibile, che il Governo ci dicesse che cosa ha intenzione di fare di questo provvedimento, perché sappiate - e i colleghi Capigruppo me ne sono testimoni che nell'ultima riunione dei Capigruppo, in presenza del Presidente del Senato, il Governo ha detto: noi oggi faremo una riunione di maggioranza, ma questi temi non interesseranno non interesseranno il Senato, perché tanto gli emendamenti verranno fatti alla Camera. E meno male che all'ultima riforma costituzionale avete votato per il bicameralismo parlamentare,

E soprattutto - mi rivolgo ancora al Governo - se non ci ritenete troppo indiscreti, se non violiamo la vostra *privacy* di maggioranza, potremmo sapere quali sono gli emendamenti che avete intenzione di presentare alla Camera

che non solo la Costituzione, ma anche recentemente la Corte costituzionale vi ha chiesto di rispettare. Rispetto gli accordi di maggioranza, ma quando diventano baratti sulla pelle baratti sulla pelle dei cittadini italiani non li possiamo accettare più. Anche in questo caso, colleghi, ci siamo trovati di fronte a un baratto. La scorsa settimana eravamo presenti, come parlamentari e come Uffici, abbiamo atteso che le Commissioni si riunissero e che la maggioranza ci dicesse qual era il frutto delle sue mediazioni, ma visto che la mediazione ancora non si era realizzata, abbiamo atteso invano, non noi parlamentari, ma gli italiani che ci stavano guardando, perché questi sono i nostri danti causa. Queste sono le persone a cui rispondiamo. È a loro - solo a loro - che noi dobbiamo rispondere. Ma non solamente noi, anche voi, colleghi. Ricordatevi che, anche in questo caso, non basterà fare un baratto (voi mi date

anche noi riteniamo che i relatori di minoranza debbano assistere alle sedute della Commissione bilancio. È per questo motivo che avanziamo una proposta. Non dipende da noi

da non consentire ai relatori di minoranza di dibattere all'interno della Commissione competente sull'appostamento di fondi, perché - lo vedremo, colleghi - questo provvedimento è una grande bugia,

Ritengo che la seduta debba riprendere intorno alle ore 17,30, con l'augurio che la Commissione bilancio abbia terminato i propri lavori.

Il provvedimento in esame è stato incardinato in Commissione il 30 gennaio scorso. I lavori sono stati caratterizzati da un calendario fitto di impegni, iniziati il 4 febbraio con le audizioni che si sono concluse il il 6 febbraio e che hanno contribuito a migliorare il testo, permettendoci di avere una visione più ampia dello stesso. Nello specifico, la Commissione ha audito 65 soggetti tra organizzazioni, enti e associazioni e ha inoltre acquisito nove memorie da parte di associazioni ed enti, oltre che la memoria del Garante per la protezione dei dati personali. Sono pervenuti, tra l'altro, diversi contributi da professori esperti in materia.

Alcune di queste proposte emendative riguardano la possibilità, per il disabile, di aderire al percorso di inserimento nel mondo del lavoro previsto per i percettori di reddito di cittadinanza

dagli oneri delle assicurazioni INAIL per i lavori di comunità previsti per i beneficiari di reddito di cittadinanza. accolti anche emendamenti di maggioranza e di opposizione che hanno previsto il coinvolgimento dei patronati per le richieste di pensione di cittadinanza.

alla possibilità di non perdere l'incentivo ove fosse licenziato per giusta causa il beneficiario del reddito superati i trentasei mesi dall'assunzione.

le proposte di maggioranza che quelle di opposizione - dà la possibilità ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di stipulare il patto di formazione attraverso specifici avvisi pubblici, previa intesa

Quello che stiamo per discutere è un provvedimento unico, doveroso e necessario per salvaguardare la coesione sociale in questo Paese. *(Applausi che tanti altri Paesi hanno messo da tempo in atto, una misura che viene proprio dall'esigenza di contrastare una situazione aggravatasi negli anni e precipitata durante la crisi economica internazionale che ha portato l'Italia a possedere il non invidiabile *record* del più alto tasso di incremento dei soggetti a rischio di esclusione sociale un dato statistico che, di fatto, si tramuta in milioni di persone in povertà assoluta e una decina di milioni in povertà relativa. L'urgenza del provvedimento è confermata dai dati ISTAT. Secondo la più recente indagine dell'Istituto nazionale di statistica sulla povertà in Italia, le famiglie in povertà assoluta sono oltre 1.700.000 e al loro interno vivono circa cinque milioni di individui. Il provvedimento è necessario anche alla luce del Pilastro europeo dei diritti sociali che all'articolo 14 prevede, e lo scandisco, che: «chiunque non disponga di risorse sufficienti, ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l'accesso a beni e servizi».

reintegrazione nel mercato del lavoro». Proprio queste sono *ratio* e finalità del reddito di cittadinanza. Ed è proprio l'articolo 1 del provvedimento che definisce in modo inequivocabile l'obiettivo della misura che ridefinisce il modello di benessere collettivo adottato fino ad ora dallo Stato italiano, abbandonando per sempre l'attuale organizzazione frammentaria e indirizzando le scelte politiche verso l'adozione di un sistema volto a ridurre l'esclusione sociale e ad accrescere la possibilità di sviluppo di ciascun individuo nell'ambito della moderna società organizzata. I meccanismi attraverso cui realizzare tale obiettivo vanno ricondotti dunque a una misura unica fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione, attraverso politiche dirette al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di marginalità, nella società e nel mondo del lavoro, in piena attuazione dell'articolo 38 della nostra Costituzione. Dunque una misura di sostegno al reddito, ma non solo, una misura proattiva, un grande investimento nei centri per l'impiego, nell'interoperabilità delle banche dati e nelle politiche attive del lavoro. Chi sono i beneficiari del reddito di cittadinanza? Si tratta di nuclei familiari che sotto il profilo del reddito e del patrimonio possiedono un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 9.360 euro; un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro; un valore del patrimonio mobiliare fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo e di 5.000 euro per ogni componente con disabilità. Il beneficio economico è composto da due elementi: uno ad integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicati per uno se si tratta di un nucleo familiare formato da un solo individuo e aumentato di 0,4 per ciascun componente maggiorenne o di 0,2 per ciascun componente minorenne del nucleo familiare; l'altro elemento che compone il beneficio economico copre le spese per i beneficiari residenti in abitazione in locazione fino a un massimo di 3.360 euro annui, o per i nuclei residenti in abitazioni di proprietà per le quali è stato acceso un mutuo. Il beneficio in questo caso copre le spese fino a un massimo di 1.800 euro annui. Per comprendere meglio come è composto il beneficio e quale sarebbe il sostegno al reddito per le famiglie, vorrei portare in Assemblea alcuni esempi. Una famiglia composta da due adulti e un figlio minore percepirà un beneficio comprensivo di rimborso per le spese di affitto pari a 1.080 euro; una famiglia composta da due adulti e tre minori percepirà un beneficio comprensivo di rimborso per le spese di affitto pari a 1.280 euro; una famiglia composta da due adulti e quattro figli minori percepirà un beneficio comprensivo di rimborso per le spese di affitto pari a 1.330 euro.

È previsto infatti un sistema di condizionalità collegato al godimento del beneficio che si estrinseca nel Patto per il lavoro e nel Patto per l'inclusione sociale. Tali condizioni contengono la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, l'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale, che comprendono accanto a specifici percorsi formativi e di ricerca attiva del lavoro, anche attività di servizio per la comunità, riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inclusione sociale e all'inserimento nel mercato del lavoro. Al rispetto delle suddette condizioni sono tenuti tutti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e non frequentanti un regolare percorso di studio o di formazione. inoltre, è che da tali obblighi possono essere esonerati i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza, nel nucleo familiare, di soggetti minori di tre anni di età, ovvero con disabilità grave o non autosufficienza. A questo proposito vorrei anche spiegare all'Assemblea il motivo per il quale non sono stati accolti alcuni emendamenti, che collegavano il carico di cura ad un comma della legge di stabilità del 2017, in materia di *caregiver*. Dato che

a tale Comitato ristretto e a quello che poi la Commissione vorrà mettere in atto sulla figura del *caregiver*. Con riguardo alla nozione di offerta di lavoro congrua, si fa rinvio ai criteri posti dal decreto ministeriale

che in verità è stata in parte modificata, in quanto il decreto ministeriale sull'offerta di lavoro congrua faceva riferimento cento in più rispetto all'ultima NASPI percepita dal beneficiario. Essendo però, in questo caso, il beneficiario del reddito di cittadinanza non un beneficiario di NASPI e cambiando la normativa, abbiamo ritenuto opportuno accogliere l'emendamento in tal senso, riguardante la retribuzione congrua. Nello specifico, la distanza dell'offerta di lavoro dal luogo di residenza, invece, è incrementata fino a comprendere l'intero territorio nazionale al crescere

ai fini della valutazione della congruità della distanza rileva anche la circostanza che nel nucleo familiare siano presenti o no componenti con disabilità. Anche in questo caso, come dicevo all'inizio, sono state apportate delle modifiche di maggior favore per le famiglie che, all'interno, hanno componenti con disabilità. Come incentivo all'immediata occupabilità del beneficiario si prevede che, qualora sia accettata un'offerta relativa ad un luogo di lavoro situato ad oltre 250 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il reddito di cittadinanza, a titolo di compensazione delle spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego, elevati a dodici mesi nel caso in cui siano presenti nel nucleo familiare componenti di minore età, ovvero componenti con disabilità. Per quanto concerne la richiesta, il riconoscimento e l'erogazione del beneficio, quest'ultimo può essere chiesto presso gli uffici di Poste Italiane o mediante un canale telematico o presso un centro di assistenza fiscale. Il riconoscimento da parte dell'INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda al medesimo INPS. Il beneficio viene attribuito mediante una carta, la quale consente, oltre che il soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, di effettuare prelievi in contante entro un limite mensile pari a 100 euro per singolo individuo, che invece viene moltiplicato per la suddetta scala di equivalenza per i nuclei con più di un componente, nonché di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione o dell'intermediario che ha concesso il mutuo. È altresì previsto che ai beneficiari del reddito di cittadinanza si applichino le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate. Il reddito di cittadinanza costituisce, tra l'altro, un importante investimento nell'interoperabilità delle banche dati, nei centri per l'impiego e nelle politiche attive del lavoro. L'articolo 6 si occupa, infatti, dell'interoperabilità delle banche dati, cioè della creazione di un sistema informativo unico in grado di collegare tutte le informazioni inerenti il lavoro e il lavoratore e un sistema nazionale per l'incrocio di domanda e offerta di lavoro che sia punto di riferimento per cittadini, imprese ed operatori del settore. Nello specifico, per quanto concerne l'attivazione e la gestione del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, è prevista l'istituzione di due apposite piattaforme digitali dedicate al reddito di cittadinanza: il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro per il coordinamento dei centri per l'impiego e il Sistema informativo unitario dei servizi sociali per il coordinamento dei Comuni. Le suddette piattaforme rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni sia tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia, nell'ambito dei servizi territoriali, tra i centri per l'impiego e i servizi sociali. Altre disposizioni riguardano le modalità operative delle citate piattaforme che costituiranno il portale delle comunicazioni dai centri per l'impiego, dai soggetti accreditati e dai Comuni all'ANPAL, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'INPS. Centrali nell'impianto del provvedimento risultano l'apparato sanzionatorio e il sistema di incentivi dedicati a imprese, enti di formazione accreditati e beneficiari di reddito di cittadinanza che intraprendono percorsi di autoimprenditorialità. Per quanto concerne le sanzioni, vengono stabilite cause di revoca o decadenza dal reddito di cittadinanza, ovvero di riduzione del medesimo, e alcune sanzioni penali in materia, oltre a prevedere specifici obblighi di comunicazione e di controllo da parte di pubbliche amministrazioni. Sono previsti inoltre incentivi in favore dei datori di lavoro privati che assumano, a tempo pieno e indeterminato, soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza; degli enti di formazione accreditati, qualora essi concorrano all'assunzione dei suddetti beneficiari; dei beneficiari medesimi che avviino un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del reddito di cittadinanza. L'incentivo per il datore di lavoro consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore, fino ad un massimo di 780 euro mensili, per un periodo non inferiore a cinque mensilità e pari alla differenza tra diciotto mensilità e quello già goduto; tuttavia, qualora l'assunzione concerna un soggetto che stia godendo di un rinnovo del reddito di cittadinanza, l'esonero è attribuito nella misura fissa di cinque mensilità. Se l'assunzione è conseguente ad un percorso formativo, svolto a cura di un ente accreditato, la misura dell'incentivo è ridotta alla metà e la restante metà è attribuita all'ente di formazione nella misura massima di 390 euro.

L'incentivo in favore dei titolari del reddito di cittadinanza per le iniziative summenzionate è costituito da un beneficio ulteriore, in un'unica soluzione, pari a sei mensilità del reddito di cittadinanza, nei limiti di 780 euro mensili. Le medesime agevolazioni sono riconosciute nel rispetto della disciplina europea cosiddetta *de minimis* e sono compatibili ed aggiuntive rispetto a quelle introdotte con la legge di bilancio per il 2019, relative ad alcune assunzioni nelle Regioni del Mezzogiorno. Qualora il datore abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza di quest'ultima disposizione, gli incentivi in esame sono fruiti sotto forma di credito di imposta. Il reddito di cittadinanza costituisce quindi un ponte tra cittadini e imprese, che punta sulla formazione continua, mirata alla creazione di competenze in linea con le professionalità richieste dall'evoluzione del mercato del lavoro. Formazione continua che costituisce il cuore del percorso per il reinserimento lavorativo dei cittadini, e che garantisce l'acquisizione di nuove competenze indispensabili a consentire la transizione da un impiego ad un altro in un mercato del lavoro in costante evoluzione. circostanza permette alle imprese di affrontare la rivoluzione tecnologica in atto potendo disporre di personale qualificato. Chiudono il Capo sul reddito di cittadinanza le previsioni relative all'assegno di ricollocazione ed altro. L'attuazione del reddito di cittadinanza si stima abbia un impatto notevole sull'intera economia nazionale. La sua erogazione fornisce un forte incentivo per la componente della platea di beneficiari potenziali che si trova nella condizione di inattività a tornare attivamente alla ricerca di lavoro. Oltre all'impatto macroeconomico generato dai consumi innescati dal reddito di cittadinanza, anche gli incentivi alle imprese aumentano le probabilità di riassorbimento dei beneficiari del programma all'interno della forza lavoro, creando un aumento della domanda interna superiore agli anni precedenti. Proprio per questo, il reddito di cittadinanza si configura come uno strumento volto a perseguire una crescita non inflazionistica, grazie alla possibilità di reintrodurre lavoratori scoraggiati all'interno della forza lavoro, che si manifesta contemporaneamente allo stimolo per la domanda di breve periodo. In quest'ottica, il potenziamento dei centri per l'impiego costituisce una vera e propria riforma strutturale. Esperienze di politiche attive praticate nei Paesi dell'Unione europea, come la Germania, mostrano come l'attivazione permanente di categorie di lavoratori precedentemente estranei alla ricerca attiva di lavoro abbia effetti sul tasso di partecipazione tali da rendere tali da rendere le politiche di inclusione attiva non soltanto stimoli positivi della domanda di breve periodo, ma anche strumenti capaci di produrre effetti sulla crescita potenziale. Con tale provvedimento gettiamo le basi per un nuovo Stato sociale, realizzando un nuovo statuto delle garanzie, non solo del lavoro, ma del concetto stesso di cittadini; un concetto idoneo a ridisegnare il diritto all'esistenza e a garantire una piena autodeterminazione dei cittadini. Concludo - e poi cedo la parola alla relatrice, senatrice Nisini, per la relazione ringraziando alcuni dei parlamentari che nella scorsa legislatura sono stati con me in questo percorso, tutti i parlamentari del MoVimento 5 Stelle, il presidente Daniele Pesco, che ha contribuito insieme a me

che introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, il diritto a conseguire la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a sessantadue anni e di un'anzianità contributiva minima di trentotto anni (la cosiddetta quota 100). La possibilità viene ammessa in favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, nonché in favore degli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche dell'INPS. II comma 1 specifica che il diritto alla pensione in base alla nuova fattispecie, conseguito entro il 31 dicembre 2021, può essere esercitato anche successivamente a tale data ed esclude che il relativo requisito anagrafico sia successivamente adeguato secondo la disciplina relativa agli elevamenti di determinati requisiti pensionistici in base agli incrementi della speranza di vita. Da tale esclusione consegue che anche nel 2021, cioè nell'anno finale del triennio interessato dal nuovo istituto, il suddetto requisito anagrafico resterà pari a Il comma 3 prevede che la pensione anticipata in oggetto non sia cumulabile, dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Vorrei soffermarmi brevemente sull'emendamento 14.27, approvato dall'11a Commissione in sede referente, che propone, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dall'applicazione del presente articolo 14 sul sistema scolastico e di garantire lo svolgimento dell'attività didattica, che nel primo dei concorsi pubblici per docente nella scuola secondaria, bandito secondo le ordinarie procedure successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le graduatorie di merito siano predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al 40 per cento di quello complessivo e che al servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione (scuole pubbliche e scuole paritarie paritarie private) sia attribuito un punteggio fino al 50 per cento di quello attribuibile ai titoli. L'articolo 15 concerne, invece, la disciplina generale della pensione anticipata, consistente in un'anzianità contributiva di quarantadue anni e dieci mesi per gli uomini e quarantuno anni e dieci mesi per le donne, e introduce un termine dilatorio di decorrenza del trattamento. L'articolo 16 dispone una proroga dell'istituto cosiddetto «opzione donna». Il nuovo intervento consente alle lavoratrici nate entro il 31 dicembre 1960 ovvero nate entro il 31 dicembre 1959, se lavoratrici autonome - di accedere alla pensione anticipata con trentacinque anni di contribuzione, a condizione che sia esercitata l'opzione per il sistema di calcolo contributivo integrale. L'articolo 17 concerne i requisiti per la pensione anticipata in favore dei cosiddetti lavoratori precoci. L'articolo 18 proroga dal 2018 al 2019 l'applicazione dell'istituto sperimentale dell'APE sociale, costituita da un'indennità pre-pensionistica in favore di soggetti aventi determinati requisiti contributivi e anagrafici rientranti in almeno una tra specifiche fattispecie, inerenti alla sfera personale o familiare o lavorativa. L'articolo l8-*bis* - proposto dall'emendamento 18.0.1, approvato dall'11a Commissione in sede referente - dispone la sospensione del pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia o anticipati, erogati dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, per alcuni soggetti condannati che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena nonché per i soggetti evasi o latitanti. L'articolo 19 sospende fino al 31 dicembre 2021 i termini di prescrizione per il pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei contributi previdenziali dovuti per i propri dipendenti per i periodi di competenza precedenti il 1° gennaio 2015. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore. I commi da 1 a 5 dell'articolo 20 introducono, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, per alcuni soggetti rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale, la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria, a condizione che tali periodi siano compresi tra la data del primo contributo e quella dell'ultimo contributo comunque accreditati. L'articolo 21 introduce la possibilità, per alcuni dipendenti pubblici, di escludere l'applicazione del limite massimo di imponibile contributivo e di base di calcolo del trattamento pensionistico. I commi 1 e 2 dell'articolo 22 introducono la possibilità di una nuova tipologia di trattamento a carico dei fondi di solidarietà bilaterali, consistente in un assegno straordinario in attesa del conseguimento dei requisiti per la pensione anticipata di cui al precedente articolo 14 (la cosiddetta quota 100). Il comma 1 dell'articolo 23 prevede che i termini temporali per la corresponsione del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici che accedono al pensionamento anticipato ai sensi del precedente articolo 14 decorrono dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata di cui all'articolo 24. Mi soffermo velocemente sull'emendamento 23.11, il quale propone di specificare che la normativa riguarda anche i soggetti che abbiano avuto accesso ai suddetti pensionamenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Secondo il testo del decreto-legge, il limite massimo della somma concedibile è pari a 30.000 euro, ovvero è pari all'importo spettante al personale che richiede il finanziamento, ove l'indennità di fine servizio, comunque denominata, sia inferiore. L'emendamento 23.21 propone di elevare a 45.000 euro l'importo massimo, fermo restando il limite concorrente, costituito dall'importo dell'indennità medesima; il medesimo emendamento prevede che l'eventuale quota ulteriore, derivante dal suddetto elevamento, possa essere chiesta anche dai soggetti che abbiano già presentato la domanda di finanziamento. Infine, l'articolo 24 riduce l'aliquota IRPEF sull'indennità di fine servizio per i casi in cui la corresponsione avvenga oltre i dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. L'emendamento 24.8 propone l'introduzione di un comma 2-*bis*. Tale disposizione consente ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che mantengano il trattamento di fine servizio, comunque denominato presso il proprio bilancio, di ottenere l'erogazione dello stesso entro novanta giorni dalla data di cessazione

esame consta, in realtà, di due provvedimenti (reddito di cittadinanza e quota 100), che poco hanno a che fare l'uno con l'altro. Ma tant'è, abbiamo capito tutti che devono essere approvati contemporaneamente e il più presto possibile, perché solo così la maggioranza può stare in piedi, anzi - mi correggo - seduta sulle proprie poltrone. *(Applausi Il reddito di cittadinanza è una bandiera del MoVimento 5 stelle, mentre la Lega contribuisce con la parte che riguarda quota 100. Ora, essendo il reddito di cittadinanza da anni, anzi da sempre, un cavallo di battaglia dei pentastellati, ci saremmo aspettati già dall'inizio dei lavori una proposta strutturata, completa, definita. Invece, abbiamo dovuto constatare, in Commissione in sede referente, che le idee su come realizzare gli *slogan* ripetuti in campagna elettorale erano poche e

o perché in attesa delle consultazioni della "magica" piattaforma Rousseau. Di questo siamo stati ostaggio. *(Applausi dal Gruppo l'articolo 1 definisce il reddito di cittadinanza quale misura a garanzia del diritto del lavoro e, nello stesso tempo, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale. Per chi ha un'età pari o superiore a sessantasette anni il reddito di cittadinanza assume la denominazione di pensione di cittadinanza. Ma, così com'è realizzato, il reddito di cittadinanza rappresenta una misura meramente assistenzialistica, solo questo, e lo vedremo. L'articolo 2 definisce i beneficiari del reddito. La platea dei beneficiari dai quasi 6 milioni di poveri promessi in campagna elettorale è ristretta a circa 1,3 milioni tra singoli e nuclei familiari a causa delle insufficienti, anche se assai cospicue, risorse a disposizione.

che c'è un tetto massimo, alla scala di equivalenza e, quindi, le famiglie numerose non sono avvantaggiate. Ciò è tanto vero che il primo effetto scaturito è stato un aumento clamoroso delle separazioni, per cui si è dovuto inserire un emendamento *ad hoc* per controllare i cambi di residenza ai fini del reddito. Peccato però - e lo voglio ricordare - che i controlli dei cambi di residenza esistono già, per cui nulla di nuovo, nulla. Sono ignorati i disabili e le famiglie che li accudiscono: le loro indennità di accompagnamento o altre forme assistenziali contribuiscono a costituire il reddito ai fini ISEE, invece di essere considerate come esigenze intrinseche alla loro disabilità. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Lo strumento «reddito di cittadinanza» si rivolge, oltre che ai cittadini italiani, anche ai cittadini dei Paesi dell'Unione europea, agli extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo. La Lega ha proposto un emendamento per circoscrivere la platea dei beneficiari extracomunitari, ma si tratta di un controllo di propaganda solo apparentemente stringente. Da questo vincolo, infatti, sono esclusi quei Paesi in cui la documentazione richiesta non è ottenibile. Quindi, gli extracomunitari provenienti da Paesi tipo Nigeria o Ecuador godranno comunque del reddito di cittadinanza, diversamente dai cittadini italiani ed europei sottoposti alla totalità dei vincoli previsti. Vi ricordo

risultano complessi e farraginosi, coinvolgendo diversi soggetti tra enti locali, INPS, INAIL, CAF, centri per l'impiego e così via, come ampiamente illustrato negli articoli 4, 5 e 6. Peccato - e questo è gravissimo - che nulla sia pronto per prendere in carico il beneficiario al momento dell'erogazione del reddito a partire dal 1°

così come i contratti di collaborazione per i 6.000 *navigator* presso ANPAL Servizi spa, da dislocare poi nei centri per l'impiego che rappresentano delle articolazioni delle Regioni che non sono state ascoltate. paradossalmente sarà erogato senza che il beneficiario possa essere preso in carico: assistenzialismo puro e tutti sanno, a cominciare dalla maggioranza, che questa situazione si protrarrà per forza di cose per molto tempo ancora. Il reddito di cittadinanza può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. Non c'è peraltro limite alla rinnovabilità, il che certifica, appunto, la consapevolezza del Governo che lo schema di proposte di lavoro definito dalla norma è semplicemente irrealizzabile. Quindi, il reddito di cittadinanza si limiterà a essere una mera erogazione economica nel più puro stile assistenzialistico, favorendo oltremodo il lavoro in nero e i controlli non saranno certo sufficienti a debellare i furbetti con una platea di beneficiari così vasta: tutto ciò finché le risorse non saranno esaurite. Le Regioni lamentano - e lo hanno fatto ufficialmente in sede di audizione - di non essere state coinvolte per quanto attiene alle loro competenze per il provvedimento, tantomeno i Comuni, che dovranno mettere a disposizione i servizi sociali e tutta l'attività amministrativa.

dovendo per di più gestire sui territori un malcontento generato dalle false aspettative prodotte da questo Governo. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Un altro aspetto di criticità riguarda la *privacy* dei richiedenti e delle loro famiglie. Come sottolineato anche dal Garante per la protezione dei dati personali*,* l'intero meccanismo non assicura la tutela dei trattamenti su larga scala dei dati personali e non appare dunque idoneo a soddisfare i requisiti richiesti dal regolamento europeo. un problema di vasta portata, che le norme vigenti imporrebbero di risolvere in tempi strettissimi, ma che il Governo ha ignorato. L'articolo 8 del provvedimento ha un titolo evocativo: «Incentivi per le imprese e per il lavoratore». In realtà esso prevede ben poche agevolazioni per i datori di lavoro, innanzitutto perché riguardano solo le aziende che hanno intenzione di fare assunzioni a tempo indeterminato Si restringono così le opportunità occupazionali dei percettori di reddito di cittadinanza, lasciando fuori tra l'altro un comparto importante che voi avete sempre trascurato in questa legislatura, e cioè quello stagionale dell'agricoltura e del turismo. Inoltre, il provvedimento prevede esclusivamente la possibilità di detrarre parte dei contributi previdenziali per un periodo troppo breve e contempla sanzioni nel caso di licenziamento entro

oltre a sottoscrivere al momento dell'assunzione del beneficiario un patto di formazione o di riqualificazione professionale? Noi abbiamo qualche dubbio e si rischia di ripetere precedenti esperienze di incentivi per i datori di lavoro assolutamente inefficaci e inutilizzate. Signori, prima di distribuirli, bisogna far sì che i posti di lavoro vengano creati. Ci vuole ben altro per creare i posti di lavoro: bisogna attivarsi per diminuire le tasse e la burocrazia, intervenire sul cuneo fiscale, creare infrastrutture, la TAV *in primis*. rendere competitive le nostre imprese con quelle straniere, attivare accordi con i Paesi stranieri per incrementare l'*export.* Solo così si crea lavoro, non solo con piccoli sgravi contributivi, oltretutto a rischio penale.

di 6 milioni di poveri, poi di 2,2, ora si parla di 1,3 milioni di nuclei familiari, mentre prima ho sentito parlare di 1,7 milioni. Sono numeri in libertà, senza contare che la formazione per i percettori di reddito costa e non si sa chi la pagherà:

ben oltre la recessione tecnica che stiamo vivendo - c'è quindi un rischio concreto che si riveli una misura solo temporanea che lascerà i poveri ancora più poveri una volta bloccata l'erogazione del reddito.

la riduzione dei requisiti di anzianità contributiva per il pensionamento anticipato, il blocco fino al 2026 dell'adeguamento alla speranza di vita sia di questi requisiti sia di quelli previsti per l'accesso alla pensione anticipata dei lavoratori precoci e la proroga di un anno delle cosiddette opzione donna e APE sociale. Le disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno sessantadue anni di età e trentotto anni di contributi sono solo in via sperimentale per il triennio 2019-2021: teniamolo bene a mente. È, quindi, un provvedimento circoscritto nel tempo e nella forma e in ogni caso avvantaggia un numero relativamente limitato di italiani. Quota 100 è una semplice deroga alle regole di pensionamento, un'ennesima finestra che lascia nuovamente fuori ancora molti esodati, esclusi dopo l'ultima salvaguardia anche dalla cosiddetta legge Fornero, adottata nella scorsa legislatura e contro la quale l'attuale maggioranza aveva tuonato in campagna elettorale. Nel nostro programma di centrodestra l'argomento pensioni era ed è uno dei punti cardine, non al ribasso come si sta facendo ora, ma concepito nell'ambito di una vera e più compiuta riforma globale del sistema pensionistico, sostenuta e ripeto sostenuta - da una reale politica di investimenti per il mercato del lavoro e il settore economico nel suo complesso. Inoltre, secondo il comma 3 dell'articolo 14 il reddito da pensione quota 100 non è cumulabile con quelli di lavoro dipendente e autonomo, escludendo - quindi - i neopensionati persino da attività che potrebbero creare posti di lavoro e gettito per le casse erariali.

Tra i benefici di quota 100 prospettati dal Governo vi sarebbe un ricambio generazionale nell'occupazione. Il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio ha invece dichiarato che, nel breve periodo, quota 100 potrebbe favorire un moderato ricambio generazionale soprattutto nel settore pubblico. Nel lungo periodo, invece, l'occupazione tanto dei giovani, quanto degli anziani dipenderà dall'efficacia delle misure di incentivo alla crescita economica implementate dal Governo. Finora questo Governo ha fatto zero. *(Applausi dal fondamentale per Forza Italia e su di esso si sono sempre basati il nostro programma e le nostre proposte. Non possiamo non evidenziare come la proposta oggi in esame sia una misura non solo limitata, ma anche costosa. Nelle valutazioni ufficiali tutte le misure pensionistiche determinerebbero un aumento di spesa pari a 4,7 miliardi di euro nel 2019, 8,7 miliardi nel 2020 e 9,3 miliardi nel 2021. Ricordo che sono tutte risorse finanziate in *deficit*. Secondo le stime dell'INPS, dalle sole misure di quota 100 e di blocco degli adeguamenti alla speranza di vita per le pensioni anticipate deriverebbe un aumento del debito implicito del sistema pensionistico pari a circa 38 miliardi di euro, interamente a carico delle future generazioni.

in materia di giochi, il cui aumento fiscale è finalizzato a parte della copertura di questa misura. Ciò rivela una contraddizione intrinseca: da un lato, mettete in difficoltà questo comparto con l'aumento delle tasse; dall'altro, lo utilizzate per finanziare i vostri provvedimenti. Quindi, colleghi della maggioranza, ancora una volta mettetevi d'accordo non solo tra di voi, ma anche con voi stessi. Riassumendo, il provvedimento in esame è caratterizzato da un miscuglio di assistenzialismo e politiche attive che favorisce - da una parte - il divano per chi non ha voglia di lavorare e - dall'altra - il lavoro nero per chi vuole e può lavorare e - dall'altra ancora - la mancanza di offerte di lavoro perché il mercato è fermo. una misura limitata che non prevede il superamento della cosiddetta legge Fornero, ma costituisce l'ennesima finestra pensata per alcuni e non per tutti. Non ci si preoccupa inoltre dei giovani, sui quali ricadrà l'intero costo

Governo, colleghe senatrici, colleghi senatori, tutte le audizioni effettuate dalla Commissione lavoro sul decreto-legge in esame, pur nella consueta diversità di accenti e interessi, hanno sollevato forti dubbi sia sul disegno complessivo sia sui dettagli attuativi del provvedimento. Nonostante il coro di critiche, la Commissione ha esaminato e approvato il decreto-legge senza tenere in alcun conto le osservazioni dei soggetti auditi e respingendo tutti gli emendamenti dei Gruppi di opposizione, e sottolineo tutti perché si è ancora una volta svilito il ruolo dei parlamentari di minoranza e maggioranza. Ma vediamo i cardini del decreto-legge, le critiche avanzate in Commissione dal Gruppo del Partito Democratico e le nostre conseguenti proposte alternative che riproporremo in Aula. Reddito di cittadinanza e interventi sulle pensioni non arrivano da Marte: vanno letti all'interno di una politica economica irresponsabile, che purtroppo sta già dispiegando i suoi effetti recessivi per l'aumento dell'incertezza, il taglio degli investimenti, il deterioramento delle aspettative di famiglie e imprese. Questo decreto-legge nasce per spendere, in maniera frettolosa più che urgente, le misure ingenti stanziate nell'ultima legge di bilancio su tali provvedimenti. Parliamo di 17 miliardi sul reddito di cittadinanza, aggiuntivi rispetto ai fondi dei Governi Renzi e Gentiloni Silveri per il contrasto alla povertà, e di 21 miliardi in tre anni per gli anticipi pensionistici. Si tratta di risorse ingenti con effetti nulli, se non negativi nel caso dei prepensionamenti, sulla crescita potenziale dell'economia italiana, e con effetti redistributivi fortemente iniqui, soprattutto nel caso delle pensioni. Il problema iniziale è che le risorse sono finte in due diverse accezioni: in primo luogo, sono solo nominalmente finanziate da aumenti della pressione fiscale a partire dal 2020, da nuove clausole di salvaguardia su IVA e accise che il Governo ha già detto più volte di non voler far scattare sul serio. In secondo luogo, sono finte perché finanziano interventi che, nel caso delle pensioni, sono temporanei nella loro durata e, quindi, destinati a creare forti pressioni per ulteriori spese una volta scaduti. Se si considerano gli impegni di spesa per il 2020 e il 2021, se si guarda alle clausole di salvaguardia aggiuntive contenute nella legge di bilancio, il 48 per cento dei soldi pubblici che nel 2020 e nel 2021 copriranno gli interventi che stiamo discutendo in questa sede semplicemente non esiste. Un euro ogni due è una finzione contabile. Quei soldi andranno trovati nella prossima legge di bilancio nel mezzo di una recessione e con nuove promesse e nuove spese da accomodare. Auguri! Rispetto al secondo punto, la temporaneità degli interventi, le risorse sono finte perché la bomba a orologeria che si sta piazzando sotto la possibilità di onorare in futuro i diritti previdenziali e assistenziali degli italiani è sconcertante.

Ma soprattutto quota 100 non è una riforma strutturale, perché è introdotta per soli tre anni. Non c'è alcun superamento della riforma Fornero: c'è solo l'ennesimo canale frammentato e temporaneo di accesso alla pensione anticipata. Non è neanche una finestra, non è un intervento tampone: quota 100 è semplicemente una lotteria. Se maturi i requisiti richiesti da qui alla fine del 2021, fai bingo; altrimenti arrivederci e grazie. Pensiamo a due persone che hanno iniziato a lavorare lo stesso giorno e hanno maturato esattamente gli stessi anni di contributi nella loro vita. Entrambi raggiungeranno l'agognata quota di trentotto anni di contributi nel 2021, ma la prima

e soprattutto se sia sostenibile politicamente. Non c'è bisogno di essere degli indovini per capire che cosa un politico, nella pienezza delle proprie facoltà, farà nell'autunno del 2021, in piena legge di bilancio, di fronte alle richieste della seconda persona di andare anch'essa in pensione a sessantadue anni, come la prima.

Altro che superamento della riforma Fornero: con queste scelte irresponsabili si prepara il terreno per una «Fornero due, la vendetta», una riforma ancora più dura, dettata - anche questa volta - dall'irresponsabilità di chi l'ha preceduta. Vediamo ora a chi andranno i benefici della lotteria, a chi andranno i benefici dei 21 miliardi spesi nei prossimi tre anni. I vincitori - come hanno spiegato tutti gli osservatori indipendenti nelle audizioni - sono persone che rispondono a un *identikit* ben preciso; sono lavoratori maschi che hanno storie contributive più robuste e hanno maturato pensioni molto più alte della media. Non solo: quelli che riceveranno il premio maggiore hanno pensioni calcolate in larga parte sul metodo retributivo. Avevano quindi già vinto la lotteria nel la cosiddetta riforma Dini, quando sono stati esclusi anche col proquota dal calcolo contributivo, e adesso avranno un nuovo premio. Insomma, sono i soliti noti del *welfare* all'italiana: non i più deboli, ma categorie elettoralmente ben rappresentate e robuste. Tra loro, stando alle prime domande delle ultime settimane, sono sopra rappresentati i dipendenti pubblici, ponendo problemi aggiuntivi di funzionamento della macchina pubblica a fronte di flussi di prepensionamento non programmati, senza che ci siano né risorse certe, né il superamento dei limiti alle assunzioni, da ultimi quelli che avete esteso nell'ultima legge di bilancio per poterli rimpiazzare. Dalla scuola alla sanità c'è un pezzo dello Stato italiano deputato a erogare servizi messo a rischio dall'incapacità di programmare e di prevedere detti prepensionamenti, anche con buona pace della propaganda sulla sostituzione tra lavoratori che escono e assunzioni di giovani. Chi pagherà il costo di questa lotteria? Lo pagheranno tutti i pensionati con assegni superiori a tre volte il minimo, a cui siete tornati a mettere le mani in tasca, più di un miliardo all'anno nei prossimi anni; lo pagheranno i giovani per cui il decreto-legge non fa niente, se non mettere a rischio l'adeguatezza delle loro pensioni future. Lo pagheranno anche le categorie più deboli

Si continua a usare, rispetto al tema dei prepensionamenti, la retorica e spesso anche l'esempio di un problema reale, vissuto da persone in carne e ossa, di un lavoratore edile che a sessantadue anni deve ancora salire su un'impalcatura.

che va oltre i trentotto anni di contributi. Lo stesso discorso vale per chi si prende cura di familiari e persone con disabilità. Per questo nei nostri emendamenti proponevano di usare una parte di quelle risorse per fare quota 92, e non 100, ma non per tutti; non per i soliti noti del *welfare* italiano, perché non tutte le condizioni sono uguali, non tutti i lavori sono uguali, e la politica ha la responsabilità di distinguere e fare delle scelte. Per tale ragione proponevamo di usare 3 miliardi del fondo per disoccupati, lavoratori in occupazioni gravose e usuranti, persone con disabilità o familiari che si prendono cura di persone con disabilità. Questo avrebbe permesso di mettere al centro le persone con condizioni di bisogno e in difficoltà e di lasciare una parte delle risorse per la crescita, gli investimenti e il taglio del costo del lavoro.

opzione donna, fino al 2022, per poi farla convergere verso una nuova e più equa flessibilità in uscita, e una pensione contributiva di garanzia per i giovani che non hanno certezza dell'adeguatezza delle loro pensioni, se hanno carriere discontinue o redditi bassi nel sistema contributivo. Invece della lotteria di quota 100 per i soliti noti del *welfare* italiano, si sarebbe potuto fare di più, a partire dalle persone in condizioni di bisogno, dalle donne e dai giovani,

il reddito di cittadinanza. In questo caso c'è poco da aggiungere rispetto all'analisi fatta dall'Alleanza contro la povertà, un grande esempio di *partnership* del sindacato e del terzo settore,

per il contrasto alla povertà nel Paese - ma peggiori risposte. Il rischio è che queste peggiori risposte finiscano per mettere a rischio, fra pochi anni, anche le maggiori risorse, quando le aspettative che si sono create verranno disattese. Quella in esame è una misura ibrida, che vuole prendersi cura della lotta alla povertà e anche favorire il lavoro, ma lo fa in maniera confusa, con strumenti ibridi che si sovrappongono tra di loro. Questa non è solo una critica "in punta di disegno", ma è una critica che mette in evidenza come il fatto di cercare continuamente di portare a casa troppi obiettivi con lo stesso strumento finisca per lasciare indietro proprio le persone che non devono essere lasciate indietro. sul reddito di cittadinanza è pieno di "invisibili", che si aspettano tanto da un passo avanti del nostro sistema di *welfare* nel contrasto alla povertà, ma che non troveranno risposte adeguate per come è disegnato l'intervento. Sono invisibili i minori e le famiglie numerose. Lo hanno detto tutti: c'è una scala di equivalenza mai vista. Il 53 per cento dei percettori di reddito di inclusione era costituito da famiglie con minori, mentre solo il 27

componente. Non ci sono servizi, non c'è un'attenzione particolare per le famiglie con minori e non si aggredisce la povertà minorile ed educativa, che è la più terribile di tutte le disuguaglianze, perché è quella che si trasferisce di generazione in generazione. Sono invisibili le persone con disabilità: non c'è alcun riconoscimento dei bisogni soggettivi aggiuntivi rispetto al mero reddito delle famiglie con a carico persone con disabilità. Non c'è alcun aumento delle pensioni e degli assegni di invalidità civile, che era stato promesso nella propaganda precedente al provvedimento in esame. Ma, oltre al danno c'è la beffa, perché, in deroga a molte sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, il parametro di reddito per accedere al reddito di cittadinanza si includono anche le pensioni di invalidità sottoposte alla prova dei mezzi. I nostri emendamenti volevano superare questo aspetto, dare un maggiore riconoscimento alle famiglie con disabilità

si toglie l'assegno di ricollocazione, che deve servire a un disoccupato per avere servizi intensivi e per ritrovare subito un lavoro, per darlo ai beneficiari di reddito di cittadinanza, anche se tutti ci hanno spiegato che solo un terzo di tale platea è immediatamente occupabile con servizi di ricollocazione. Inoltre, con queste risorse si sarebbe tranquillamente raddoppiare il reddito di inclusione dal Gruppo PD)*, allargare la platea, rafforzare l'infrastruttura dei servizi e avere un residuo di 2 miliardi di euro, per dare garanzia del reddito ai disoccupati.

anche se non sono sotto la soglia di povertà e non passano una prova dei mezzi. Con i due miliardi si sarebbe potuto rafforzare il sussidio di disoccupazione allargandolo; già è stato fatto nella scorsa legislatura e adesso dura due anni invece che uno, e raggiunge il 97 dei disoccupati; ma la garanzia del reddito può essere rafforzata soprattutto per quei lavoratori con più di cinquant'anni, per i quali è difficile dare servizi di ricollocazione e formazione. Non solo, ma sono invisibili in questo provvedimento anche le persone senza fissa dimora, gli stranieri che hanno lavorato e hanno regolarmente dato un contributo all'economia italiana, gli italiani che rientrano da esperienze all'estero, magari per farsi carico di nuovi progetti di vita in Italia.

È invisibile il terzo settore, che è tutta la rete di persone che hanno lavorato in trincea per anni, da sole, nel contrasto alla povertà e si vedono scavalcate da un'infrastruttura di servizi che punta non su una presa in carico dei Comuni e del terzo settore che guarda a tutte le dimensioni della povertà, non solo quella del reddito, ma su una infrastruttura solo lavoristica e su servizi al lavoro che magicamente dei *navigator* precari dall'oggi al domani dovrebbero essere in grado di fornire.

fortemente contrari: il tema delle sanzioni penali. Avete introdotto sanzioni penali per chi rende dichiarazioni

che sono vicine alla soglia di accesso al reddito di cittadinanza che farebbero meglio a rubare che non a provare ad accedere al reddito di cittadinanza. Il Governo ci ha detto che non va bene falsificare i documenti per accedere al reddito cittadinanza. È chiaro che non va bene, ma nella Patria di Cesare Beccaria un principio cardine dello Stato di diritto e della civiltà giuridica è che l'entità della pena deve essere proporzionata e commisurata all'entità del reato. Si tratta non solo di una norma punitiva che dà il senso di una visione di povertà colpevole contenuta in molte parti del provvedimento, ma è anche il sintomo di una matrice culturale che preoccupa. Potete litigare sul tunnel della TAV, ma andate d'accordo su cappi e manette, perché la visione della convivenza civile che vi tiene insieme è giustizialista, violenta e manettara. Anche su questo, la visione del Partito Democratico è molto diversa, radicalmente alternativa.

ore 16. Come lei puoi immaginare, sono molti i motivi che mi portano a non confidare in un regolare e proficuo lavoro della Commissione bilancio. Mi limito per ora - poi riprenderò nel dettaglio questi motivi -

ricordiamo oggi Fulvio Camerini, un uomo e un senatore, scomparso da poche ore, che ha fatto onore a quest'Aula. Altri potranno descrivere le doti e il *cursus honorum* di un medico e di uno scienziato che ha lasciato un'impronta decisiva nella sua Trieste e che ha avuto riconoscimenti

A me il compito di trasmettere a quest' Aula la memoria del senatore e del politico, dell'uomo di dialogo. Nel marzo del 1995 accolse subito e con entusiasmo il progetto di unire il centrosinistra sotto il simbolo dell'Ulivo. Il *tour* delle Cento città, guidato da Romano Prodi, che diede inizio a una straordinaria pagina politica, partì proprio da Trieste. Il professor Camerini era lì, alla Stazione marittima di Trieste, a battezzare quella nuova avventura che lo portò, subito dopo, nell'aprile del 1996, a entrare a Palazzo Madama, senatore eletto nel collegio del Friuli-Venezia Giulia. Non fu facile per lui decidere di candidarsi, eppure ancora ampiamente tra gli scienziati riconosciuti in Italia e all'estero; non fu facile decidere di abbandonare l'attività medico-scientifica per dedicarsi alla politica. Non aveva mai abbandonato la medicina, e la politica avrebbe potuto rappresentare per lui una situazione sconosciuta, insidiosa, difficile. Non lo fu. Anzi, al contrario, fu per lui, e per tutti i suoi elettori e i concittadini che hanno avuto la fortuna di incontrarlo e conoscerlo, una sfida vinta sin dal primo momento. Dopo un consulto con la amatissima moglie Bianca, scomparsa solo la scorsa primavera, Camerini comunicò ai segretari politici di allora del Partito Popolare e del Partito Democratico della sinistra di Trieste che avrebbe affrontato questa prova. E a chi ebbe modo di vivere quotidianamente con lui la campagna elettorale fu evidente quale fosse il suo spessore. Camerini era fatto di pasta diversa, speciale anche in questo. Batté palmo a palmo il suo collegio senatoriale, non fermandosi praticamente mai. Aveva una parola per chiunque incontrasse o lo fermasse, talvolta i suoi pazienti che gli chiedevano un consiglio o una semplice parola di conforto. Ma chi voleva parlargli erano soprattutto i cittadini, per confidargli un problema occupazionale o legato alla vita della propria città: Camerini c'era sempre e per chiunque. Non si è mai sottratto, né allora, né in seguito: mai. Ha sempre avuto un'attenzione viva e partecipata per tutti, anche per chi vi parla, fino alla fine della sua vita terrena, proponendosi con saggezza infinita e profonda onestà. Fu eletto sotto il simbolo dell'Ulivo, un simbolo e un progetto che sentiva affine alla sua natura di cattolico di sinistra. Fu un grande dispiacere e una delusione personale, una volta eletto, non trovare quel simbolo anche tra i Gruppi parlamentari della XIII legislatura. Gli anni da senatore, come quelli da professore universitario e primario, furono intensi e trascinanti per lui che scopriva la forza dell'azione politica e di quella legislativa in particolare, ma anche per tutta la comunità triestina che ebbe la possibilità di avere per un quinquennio un confronto continuo e permanente con l'attività romana del proprio senatore. Non c'era nessuna intermediazione: Non c'era nessuna intermediazione: mentre Internet stava facendo i primi passi, il senatore Camerini convocava regolarmente assemblee pubbliche per rendere conto della propria attività parlamentare, per riferire, ascoltare le critiche, i suggerimenti e le cose da fare. Tutti potevano interloquire con lui e l'azione senatoriale ha lasciato una traccia profonda nell'attività di questa Camera e in tutta la società regionale, a cominciare dal tenace e assiduo lavoro per portare in porto la legge per l'equo indennizzo dei beni abbandonati dagli esuli istriani e giuliano-dalmati,

la sua cultura, il suo metodo rigoroso e la disciplina con cui affrontava sempre le cose gli hanno consentito di diventare da subito un politico a tutto tondo. Fulvio Camerini è stato un uomo retto e giusto, un signore e un galantuomo. Con lui scompare un grande italiano e un grande triestino. Ci mancherà moltissimo, perché in tutti questi anni Camerini era diventato un punto di riferimento non solo per la comunità scientifica servita per oltre settanta anni, ma anche per quella buona politica che tutti noi dobbiamo tendere a realizzare. Grazie Grazie Fulvio e riposa in pace. Signor Presidente, non aggiungerò molto alle parole della collega che ha descritto molto bene l'uomo Camerini e la sua passione politica. Se la politica è azione civile ed è mettersi in gioco in modo disinteressato a favore dei cittadini, allora Fulvio Camerini è stato un uomo politico. Purtroppo, qualche volta la politica non è solo questo ed è per questo che forse ha continuato a dare un grande contributo al dibattito politico, pur restando fuori dalla politica.

perché conta quanto si ha ancora da dare e da dire al dibattito politico, civile e sociale del nostro Paese. Fulvio Camerini aveva ancora tante cose da dirci e da darci. Per questo penso che si possa dire che è prematuramente scomparso, perché mancherà la sua voce per la mia città, ma penso anche per tutto il tessuto sociale del nostro Paese. Ha contribuito a creare quel sistema Trieste, insieme al professor Budinich, a Panizon e a tanti miei concittadini che hanno

ha prodotto una generazione di cardiologi che sono andati in giro per l'Italia e anche all'estero. Questa è la grandezza di Camerini. Qualcuno ricorda anche la sua particolare spiccata umanità, che evidentemente era pari al suo rigore scientifico e al suo essere

Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, bene, ci siamo quasi. Con il decreto-legge in discussione stiamo per compiere un'operazione di redistribuzione della ricchezza senza precedenti nella storia della Repubblica italiana. L'idea di un reddito minimo per le fasce più deboli della popolazione ha rappresentato la proposta politica principale del MoVimento 5 Stelle fin dalla sua nascita dieci anni fa. Lo sanno bene le migliaia di attivisti che in questi anni hanno dato l'anima con i banchetti informativi per raccontare il sogno di chi ci ha creduto fin dall'inizio, dedicandovi parte della sua vita e che oggi siamo certi sarebbe orgoglioso del risultato raggiunto; un sogno che finalmente si realizza anche grazie a chi ha fatto da cassa di risonanza con la potenza della comicità e a chi per primo sei anni fa ha presentato il disegno di legge in Parlamento.

Propaganda, cari colleghi, è fingere di non vedere che la crisi è di portata mondiale e che la globalizzazione ha fallito, che la società si aspetta una via nuova che, se non sarà mediata dalla politica, produrrà nuove diseguaglianze e nuovi conflitti tra chi ha e chi non ha. Basta guardare l'andamento della povertà assoluta in Italia tra il 2005 e il 2017, anno in cui il numero di persone in povertà assoluta ha sfondato quota 5 milioni. Praticamente, nell'arco di dodici anni il loro numero è più che triplicato. C'è da chiedersi dove fossero allora i sindacati e la sinistra e soprattutto cosa hanno fatto i vecchi Governi per gli ultimi. Evidentemente niente, perché possiamo disquisire su tutto, ma i numeri sono incontrovertibili. In tale contesto di profonda crisi economica e sociale non possiamo più limitarci ad analizzare la situazione denunciandone gli effetti criminali e ingiusti. Diventa necessario passare all'azione, ponendo attenzione ai drammatici segnali che provengono dai conflitti del mondo reale. Abbiamo il dovere di guardare dritto in faccia le disuguaglianze e di intervenire per porre rimedio ai disastri causati da scelte sbagliate. Le opposizioni continuino pure nella patetica battaglia contro la nostra riforma, lanciando raccolte firme per l'abolizione del reddito di cittadinanza, marcando così sempre

che mira a favorire il diritto al lavoro attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti a rischio di emarginazione. Scopo di questa misura è dunque garantire a tutti il pieno godimento dei diritti di cittadinanza e di socialità. Entro nel vivo del dibattito rispondendo alle critiche principali che sono state mosse fin dall'inizio a questa iniziativa e che sono spinte più da motivazioni politiche che da ragioni come - per esempio - la narrazione per cui una misura di sostegno al reddito, che assicura una somma di 780 euro, possa scoraggiare la ricerca di lavori a basso salario. In sostanza, in un Paese fondato anche sull'articolo 36 della Costituzione, che sancisce il diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, non ci si preoccupa minimamente dell'esistenza di lavori a tempo pieno da poche centinaia di euro al mese, lavori da fame, ma ci si preoccupa piuttosto della compensazione del reddito di quanti vivono sotto la soglia di povertà, che invece spingerà al rialzo i salari e le condizioni lavorative. La lotta dei disoccupati francesi - per esempio - ha avuto tra le sue parole d'ordine la richiesta non solo di un'occupazione, ma anche e soprattutto di un reddito. Il bisogno di un reddito, in quanto cittadini appartenenti a una comunità, e la possibilità di essere inseriti nel mondo del lavoro sono le richieste principali che stanno alla base delle vertenze conflittuali Che dire poi della convinzione diffusa che il reddito di cittadinanza alimenterà truffe e lavoro in nero, poiché una buona parte degli italiani sarebbe costituita da disonesti che sicuramente riusciranno ad aggirare i requisiti di accesso al beneficio? Ma coloro che sono stati definiti i fannulloni del divano dove dovrebbero trovare il tempo per oziare, oppure per lavorare in nero, viste le ore che li vedranno impegnati nella formazione, nei lavori di pubblica utilità, ma anche nella ricerca del lavoro? Stigmatizziamo ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, queste condotte illecite e rassicuriamo sulle rigorose misure di controllo che sono previste dall'articolo 7 del provvedimento, tanto nei confronti di coloro che tenteranno di accedere in modo fraudolento alla misura prevedendo, oltre a ipotesi di riduzioni e di decadenza dal beneficio, addirittura la comminazione di sanzioni penali, quanto nei confronti degli operatori dei patronati e dei centri per l'impiego che si adopereranno per informare i cittadini e non per suggerire come aggirare il sistema, se non vorranno rischiare anche loro di incorrere in sanzioni disciplinari e contabili. Quindi, se la paura che alcuni potrebbero beneficiare indebitamente del reddito porta alla convinzione che è meglio lasciare tutto per come è - e quindi le cose per come stanno - allora tanto vale che aboliamo tutte le altre misure di sostegno al reddito: aboliamo l'indennità di invalidità e pure gli ammortizzatori sociali. Ma se crediamo ancora nel senso politico della parola *welfare*, allora dobbiamo impegnarci per concretizzare un provvedimento necessario e urgente, che sicuramente è perfettibile, ma che va inevitabilmente nella direzione di una società più giusta, coesa, ma soprattutto più equa.

di un grande evento. Questi due provvedimenti cambieranno il tessuto sociale della nostra Nazione e ciò mi emoziona, come ha emozionato la senatrice Campagna. Con il reddito di cittadinanza adotteremo uno strumento per il contrasto alla povertà: 5 milioni di poveri hanno chiesto l'aiuto del Governo e il Governo c'è, il Governo è presente! No, non sono calmo. Avete creato 5 milioni di poveri. Non sono calmo; sono entusiasta di questa manovra.

dipendenti e lavoratori, sequestrati da Elsa Fornero, che non gli ha permesso di andare in pensione e di vivere la propria vita da pensionati. Questa è una vergogna e noi rilanceremo con forza quota Il mio pensiero va anche a quei sindacati che per anni sono stati assenti, in particolare la CGIL, che ha dimenticato il suo ruolo di sindacato per tornare in piazza con il rivoluzionario Landini. Oggi torni, Landini, ma dov'eri quando hanno abolito l'articolo 18? Dov'eri? Oggi scendete tutti in piazza, ma questa è una manifestazione strumentale. Noi non ci faremo intimorire e andremo avanti per la nostra strada, consapevoli di fare un vero progresso di cambiamento. Noi siamo il vero progresso. Voi non siete progressisti. avete criticato perché discutiamo in maggioranza. Ma vivaddio che discutiamo, perché finalmente c'è un Governo che non prende ordini dalle letterine dell'Unione europea; c'è un Governo che discute e porta delle soluzioni, al contrario di quanto hanno fatto i signori del centrosinistra, che aspettavano le letterine dall'Unione europea gioco di parole - di chi li comandava. Oggi questo è finito, non c'è più: ci siamo solo noi, un Governo attento a quelle che sono le esigenze del popolo, quel popolo che qualcuno ha dimenticato, e soprattutto ha dimenticato e abbandonato che oggi, grazie anche al *leader* Matteo Salvini, stiamo rimettendo al centro della nostra azione politica. azione politica. Abbiamo portato degli interventi non indifferenti, come la pace contributiva, che permetterà di riscattare i periodi scoperti dalla contribuzione, fino a un massimo di cinque anni; un atto di civiltà per chi ha perso anni di lavoro. il Fondo di solidarietà, che permetterà quel ricambio generazionale che voi avete distrutto con le vostre riforme del lavoro, che avete chiamato mercato, come se i lavoratori fossero delle bestie. Si deve chiamare non mercato del lavoro, ma mondo del lavoro:

opzione donna, di passare il loro tempo in famiglia e di farne subentrare altre nel mondo del lavoro; un atto concreto per la parità dei diritti, cosa che voi avete sempre blaterato - sì, blaterato, voglio usare questo termine - ma non avete mai portato a termine; solo chiacchiere. Invece noi stiamo facendo i fatti e porteremo cambiamenti, con il reddito di cittadinanza, con quota 100, con il Governo che andrà avanti fino in fondo.

come membro dell'opposizione. Devo dire che storicamente, come persona che è all'opposizione da diverse legislature, mi sorprendo sempre davanti a due problemi reali che si trascinano da oltre dieci anni: il problema della povertà assoluta e quello della povertà relativa, che sono in crescita e in questi anni non hanno visto alcuna flessione, con nessuna misura, né con i Governi di destra, né con i Governi di sinistra, né con i Governi tecnici, né con tutta la successione dei Governi dell'ultima legislatura, e nemmeno con questo Governo. Il problema della povertà è talmente serio che finora ha potuto misurarsi e confrontarsi solo con misure transitorie; penso alla *social card*, penso agli 80 euro renziani, penso attualmente al reddito di cittadinanza. Noi ci troviamo davanti a soluzioni sbagliate per problemi veri. E chi fa le spese di tutto questo è quella popolazione che di fatto è la più fragile. Capisco benissimo che non ci sia Governo che possa ignorare il problema della povertà. Noi siamo estremamente attenti alla povertà assoluta in crescita; siamo preoccupatissimi di quella povertà relativa che oggi riguarda l'impiegato, l'infermiere, l'insegnante, la persona che una volta avremmo considerato come facente parte della classe media e che oggi stenta ad arrivare alla fine del mese. Noi siamo preoccupati davvero per l'investimento che è stato fatto in questi anni sui nostri giovani, studenti universitari, laureati, molto spesso con *master*

Noi siamo preoccupati dalla fallacia assoluta di quello che ci state proponendo. Sono oggettivamente menzogne o, se volete, bugie pietose. Ma sapete cosa diciamo noi medici? Il medico pietoso fa la piaga cancrenosa, e cioè quando a un problema vero si oppone una soluzione sbagliata,

una stagnazione tecnica che, nel giro di pochi mesi, diventerà reale. È inutile che ogni giorno - mattina, pomeriggio e notte - ci ripetiate che non metterete mano ad alcuna patrimoniale, che non ci saranno aumenti di tasse. Siamo sconvolti dall'idea di tale ingenuità,

Signor Presidente, il reddito di cittadinanza è la prova provata di come si possa fare davvero politica per il popolo. Tra battute di dubbio gusto e attacchi misti a risentimento, i destinatari di questa riforma epocale sono stati dipinti, via via, come nullafacenti, furbi o poco di buono, come se lo stato di necessità in cui versano cinque milioni di italiani sia una loro colpa. Fa specie che tanta avversione provenga proprio da sinistra e ciò non si può spiegare solo con la logica dell'antagonismo e dell'opposizione. Credo Credo che la ragione sia più profonda e risieda nella trasformazione che ha portato buona parte di questa sinistra a far propria una visione neoliberista. Il reddito di cittadinanza quale misura proattiva e non meramente assistenzialistica - come più volte esplicitato nel corso del dibattito politico, e non solo è stato oggetto di attacchi strumentali e non neutrali. Tuttavia, in assenza di verità assolute, portare in primo piano l'elemento ragionieristico rispetto a quello sociale è assolutamente sbagliato; come è sbagliato ritenere che le indicazioni e le reazioni dei mercati - leggi *lobby* e centri d'interesse - siano determinanti per le scelte economiche di una Nazione e che per tale motivo vengano prima di ogni decisione politica. Sono punti di vista, forse, ma non di sinistra. Si può pensare che la società avrà sempre una sacca di povertà, ma è inaccettabile per un politico, di destra o di sinistra,

se tutti i consociati si attivino per trovarsi o crearsi un posto di lavoro, ma non è un ragionamento che può fare un politico. Come un buon politico non può pensare che lo Stato non debba ridistribuire le risorse facendo particolare attenzione ai più deboli, dal momento che egualitarismo e giustizia sociale sono parole impresse nella nostra Costituzione. È assai strano che a sinistra ci si scagli contro le presunte politiche di non accoglienza in nome dell'imperativo etico di soccorrere e aiutare i più deboli, per poi sostenere con altrettanta veemenza che il reddito di cittadinanza quale azione di soccorso economico alla povertà è diseducativa, se non addirittura pericolosa, perché il povero con qualche soldo in tasca in più finisce con il sentirti ricco e non si attiva più come dovrebbe per uscire dalla sua condizione. Credo che Gramsci intendesse altro quando, ponendosi in contrasto con la cultura cattolica, scrisse che i poveri devono accontentarsi della loro sorte, poiché le distinzioni di classe e la distribuzione della ricchezza sono disposizioni di Dio e sarebbe empio cercare di eliminarle. È facile capire chi dovrebbe essere oggi considerato Dio, ma la lotta di classe è ormai archiviata dalla "*nouvelle gauche*" tutta pizzi e lustrini. È facile dunque ironizzare e tragicamente ridicolizzare la scelta dell'avversario politico che, in quanto tale, porterebbe con sé la presunzione dell'errore. Ma il dato di fatto incontrovertibile è che il reddito di cittadinanza è la più importante misura di contrasto alla povertà e al tempo stesso di politica attiva del lavoro degli ultimi trenta anni. A me pare, molto più banalmente, che sempre più spesso la lingua di taluni non vada di pari passo con il pensiero che il tecnicismo e il conformismo abbiano contaminato persino le idee. Visto allora che coloro che si trovano ai margini della società non sembrano più godere delle attenzioni della sinistra, non rimane che l'artificio retorico, che suona alquanto cinico, perché mentre il gramsciano Dio cattolico contemplava almeno la carità, quello della nuova sinistra non contempla neanche quella. E allora si parla di assistenzialismo per stigmatizzare l'istituto del reddito di cittadinanza, sebbene il nostro sistema di *welfare* si regga sul modello assistenziale voluto soprattutto dalla sinistra. Qualcuno disse che «se guardi il mondo con gli occhi dei più deboli, puoi fare davvero un mondo migliore per tutti». Se si smarrisce questa prospettiva, viene meno l'idea stessa di giustizia sociale, uguaglianza e redistribuzione del reddito, che è alla base di una società civile. Allora, che dire? Ci abbiamo pensato noi del MoVimento 5 Stelle a fare davvero - ma davvero! - qualcosa di sinistra.

e per tre annualità, di andare in pensione avendo un minimo di sessantadue anni di età e trentotto di contributi. I lavoratori privati che hanno raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2018 potranno ritirarsi dal lavoro già dal 1° aprile 2019. Chi raggiungerà più tardi tali requisiti potrà andare in pensione tre mesi più tardi: la finestra è dunque di tre mesi. I lavoratori pubblici, invece, avranno finestre aperte di sei mesi, con un preavviso di Grazie gli insegnanti dovranno aspettare il 28 febbraio per fare domanda di pensionamento e lasceranno il lavoro all'inizio dell'anno scolastico successivo. Tutti coloro che optano per la cosiddetta quota 100 non potranno cumulare l'assegno con redditi da lavoro superiori a 5.000 euro l'anno, fino al raggiungimento dei sessantasette Inoltre, il loro assegno pensionistico sarà più leggero, perché avranno versato meno contributi. Per favorire ulteriormente il ricambio generazionale tra lavoratori anziani e lavoratori giovani, la legge di conversione prevede inoltre lo sviluppo di una formula già esistente, ma poco utilizzata: le imprese in crisi o con esuberi possono utilizzare i fondi di solidarietà di settore

Il fondo, con oneri a carico delle imprese, paga l'anticipo pensionistico fino al raggiungimento dei requisiti per quota 100. La novità è che le imprese non devono pagare anche i contributi per gli anni mancanti alla pensione. Il provvedimento oggi in esame si è reso necessario, alla luce degli effetti distorsivi della legge Fornero nei confronti del mercato del lavoro e dell'aumento della disoccupazione giovanile. Infatti, negli ultimi anni abbiamo assistito a un progressivo allungamento dell'età pensionabile per adeguarla alla speranza di vita dei lavoratori. La legge Fornero con il tempo è diventata una diga di contenimento a un grosso bacino di lavoratori anziani che la percepiscono con sempre maggiore insofferenza, in particolare nella pubblica amministrazione, dove il blocco del *turn over* e l'aumento dell'età pensionabile hanno aumentato l'età media dei lavoratori a cinquantacinque anni, un po' troppo elevata rispetto alla media europea. Per risolvere questo problema, si è già intervenuti con il provvedimento concretezza, per sbloccare il *turn over* e consentire un rapporto di uno a uno fra lavoratori in entrata e in uscita. Quota 100 continua in questa direzione e consentirà ulteriormente il ricambio generazionale attraverso l'assunzione di giovani in sostituzione di lavoratori che andranno in pensione. Nell'arco dei prossimi tre anni, si cercherà di far defluire da questo collo di bottiglia un certo numero di lavoratori anziani, così da rendere successivamente più agevole il raggiungimento del vero obiettivo che si è posto il Governo: anni di servizio indipendentemente dall'età. Questo provvedimento sperimentale bloccherà momentaneamente l'adeguamento dell'età pensionabile alla speranza di vita e il primo scatto ci sarà soltanto nel 2021. Nel rapporto privato probabilmente non ci sarà un sicuro ricambio di uno a uno, ma si è voluto contribuire fornendo alle aziende un impulso positivo che può renderle più economiche, agili e più appetibili sul mercato del lavoro. L'opportunità di andare in pensione è stata già accolta favorevolmente da decine di migliaia di lavoratori in possesso dei requisiti e avrà un impatto positivo sul mondo del lavoro. I dati in arrivo ci consentono di dire che si può stimolare e sostenere il passaggio generazionale. Considerata l'età di molti lavoratori ancora in servizio, si può affermare che i nonni stanno lasciando il posto di lavoro ai figli, così avranno un po' di tempo da trascorrere in famiglia e con i nipotini. È altamente probabile che un posto di lavoro consenta ai nostri giovani di farsi una famiglia e favorisca anche la natalità. Quota 100 è una facoltà volontaria, un modo aggiuntivo per accedere alla pensione insieme a tutti gli altri accessi ordinari già previsti o regolati dalla riforma Monti-Fornero. Pertanto, si potrà continuare ad andare in pensione utilizzando indifferentemente sia la legge Fornero, sia quota 100, l'APE *social*, la pensione di anzianità, l'opzione donna o i provvedimenti previsti per i lavoratori precoci e quelli per le attività particolarmente usuranti. Fra le norme che stiamo approvando, si prevede anche che l'INPS effettui un monitoraggio mensile per l'anno 2019 e trimestrale negli anni seguenti sul numero delle domande di pensionamento e fornisca al Ministero del lavoro e a quello dell'economia e delle finanze la rendicontazione degli oneri che ne derivano, proprio per evitare scostamenti dalla spesa prevista. Quota 100 disciplina la riforma della *governance* dell'INPS, l'ente che gestisce le pensioni e l'assistenza, e quella dell'INAIL, l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. Essa dispone il passaggio da una gestione accentrata nelle mani dei rispettivi presidenti a una collegiale, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nei due enti verranno ripristinati i consigli di amministrazione, che erano stati aboliti molti anni prima, e saranno composti di cinque membri di nomina governativa, compreso il presidente. Relativamente all'INPS, ho maturato la personale opinione che dovrebbe essere scorporata fra assistenza e previdenza, come negli altri Paesi europei. Si farebbe finalmente luce sull'entità dei contributi versati dai lavoratori, che dovrebbero essere utilizzati esclusivamente per le loro pensioni, mentre per l'assistenza si dovrebbe provvedere con la fiscalità generale. Probabilmente, si scoprirebbe che anche gli italiani potrebbero andare in pensione molto prima dei sessantasette anni attualmente previsti dalla legge Fornero.

Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signori rappresentanti del Governo, oggi discutiamo di un provvedimento importante, che avrà per sua natura enormi ricadute sotto il profilo economico e sociale. Spesso le forze di opposizione hanno criticato la nostra misura, ritenendola assistenzialistica e non propriamente economica, ma si è resa necessaria per riportare al centro dell'attenzione e dell'azione politica i veri destinatari dei nostri lavori: i cittadini e le imprese. Vorrei soffermarmi proprio sulle imprese, in particolare su quelle piccole e medie, alle quali va il nostro ringraziamento per aver continuato a incrementare il nostro tessuto economico, nonostante le misure avverse alle quali in questi anni sono state sottoposte. Basti pensare infatti che il 56,4 per cento degli occupati del settore privato lavora in aziende con meno di 20 addetti, superando del 16,5 per cento la media europea. Proprio la tutela delle piccole e medie imprese, oltre che dei cittadini, ci ha spinto a lavorare per licenziare un provvedimento storico che possa ridare finalmente dignità a imprenditori e cittadini.

Basti pensare allo sgravio contributivo, pari alla differenza tra la durata massima del reddito di cittadinanza e le mensilità della misura già percepita al momento dell'assunzione, alle imprese che decidono di assumere a tempo indeterminato.

formazione. Diamo 780 euro non per stare stesi sul divano, come spesso ci ha rimproverato l'opposizione, ma per la formazione e l'inserimento nel mondo lavorativo. Prevediamo inoltre un contributo per gli enti di formazione accreditati che prendono in carico un beneficiario del reddito di cittadinanza per formarlo gratuitamente. Il nostro Governo e la nostra maggioranza vogliono non regalare soldi, ma fare una vera e propria riforma economica: se il beneficiario, alla fine del percorso di formazione, ottiene un lavoro coerente con il profilo formativo, i centri di formazione ottengono un beneficio pari alla metà del periodo che manca allo scadere dei diciotto mesi del reddito

per chi forma e per chi assume, facendo girare l'economia del nostro Paese, da troppi anni paralizzata da politiche di austerità dimostratesi fallimentari. Ricordo inoltre che chi percepisce il reddito ha d'obbligo, pena la perdita del beneficio stesso, di accettare una della tre proposte lavorative che gli verranno offerte. Come ho già detto, però, questa misura agevola anche l'imprenditoria. I beneficiari del reddito di cittadinanza che avviano un'impresa nei premi dodici mesi, infatti, ricevono un beneficio pari a sei mensilità del reddito. Cosa vuol dire? Vuol dire che, se un cittadino che percepisce il reddito da dieci mesi, ad esempio, avvia la propria attività, riceverà in un'unica soluzione un bonifico di 4.680 euro, pari a sei mesi del beneficio residuo, e questo per avviare la sua attività. Insomma, dopo il decreto-legge dignità, le importanti misure previste all'interno della legge di bilancio e l'approvazione del decreto-legge semplificazioni a sostegno di imprese e cittadini, con questo provvedimento andiamo ad aggiungere un importante tassello alla nuova idea di economia e società a cui aspiriamo: una società in cui si lavora per vivere e non una in cui si vive per lavorare; una società in cui ognuno abbia le stesse opportunità e gli stessi diritti; una società che ci hanno impedito di avere finora a causa di una classe politica troppo attenta ai propri interessi Incentivo alla ricerca del lavoro, avvio di attività imprenditoriali e assunzioni stabili: l'opposizione può dire che questa sia una misura assistenzialistica, ma i fatti parleranno per noi, mentre per loro hanno già parlato e verranno ricordati per aver eliminato l'articolo 18 o per aver votato la riforma Fornero. Insomma, con il Movimento al Governo le priorità sono altre: sono i cittadini e con loro le imprese, su cui dobbiamo puntare per fare in modo che la nostra economia torni a crescere. *(Applausi

colleghi, diversamente da molti di voi, sono convinta che questo sia un provvedimento che non affronta, e tantomeno risolve, Gruppo PD)*. Anzi, a me pare molto di più l'ordine di pagamento di due cambiali elettorali emesse da Lega e MoVimento 5 Stelle. Peraltro, è una proposta che - a mio avviso - tradisce le promesse annunciate: non servirà né ad abolire la povertà - «*vaste programme*» avrebbe detto De Gaulle - né a cancellare la legge Fornero. rapidamente dal reddito di cittadinanza. I costi saranno ben superiori a quelli previsti; non garantirà l'intera platea di quanti versano in condizione di povertà assoluta e, anzi, introdurrà odiose discriminazioni territoriali tra Nord e Sud, e nazionali tra cittadini italiani e cittadini stranieri. Non si istituisce una misura di sostegno universale e si postula persino l'esistenza di una rete di servizi per l'impiego, che è di fatto inesistente. Ma siete mai entrati in un centro per l'impiego?

In più, sono molto modesti - come ci ha detto l'Ufficio parlamentare di bilancio - sia le ricadute occupazionali - stiamo parlando dello 0,2 se capisco bene - sia gli effetti del reddito sul PIL (anche qui 0,2-0,4 per cento). La verità che la maggioranza e il Governo continuano a negare è che per affrontare la questione povertà sarebbe necessaria - come è stato fatto nella proposta che abbiamo avanzato come Radicali italiani - una riforma profonda e complessiva del *welfare* italiano. Aggiungere un altro istituto a quelli esistenti aumenta la spesa, ma non l'efficacia del sistema. Quindi - a mio avviso - il reddito di cittadinanza, come voi lo proponete, sarà un doppio spreco: un'occasione di riforma importante sprecata e uno spreco di ingenti risorse pubbliche. Se invece si fosse deciso di realizzare questo intervento in un arco di tempo più lungo, senza inseguire l'immediato successo elettorale, vi sarebbero state le risorse disponibili per gli investimenti più urgenti, per far crescere il Paese e più tempo per adeguare i servizi per l'impiego e i servizi sociali dei Comuni. Ma senza crescita e senza servizi efficienti - scusatemi, colleghi - gli assistiti non diventano per legge occupati. Potete fare una legge, ma questa trasformazione non avviene. Ho quasi finito il mio tempo, lo so, quindi non mi dilungherò su quota 100. Molto è già stato detto, ma - badate determinerà una discriminazione di genere importante: molte, moltissime donne, in alcune zone particolari del Paese, non hanno una carriera lavorativa continuativa. Di fatto, a beneficiarne saranno quasi esclusivamente lavoratori di sesso maschile. Si ipotizza, peraltro,

non mi sfugge che una parte della vostra fortuna sia legata alle promesse che il decreto-legge che ci accingiamo a convertire fa finta di mantenere; ma non mi sfugge neppure che l'Italia è un Paese in cui le scelte più disastrose sul piano della finanza pubblica e dell'equità sociale (non parliamo, poi, del debito pubblico) sono sempre state supportate da forti maggioranze elettorali e parlamentari: peccato che si siano rivelate disastrose. Su questo piano, non siete il Governo del cambiamento, come sostenete di essere, ma quello della continuità dei mali cronici della politica italiana, a partire dalla demagogia e dall'uso della spesa pubblica come strumento elettorale. Sareste forse potuti andare adagio, migliorando il Rei, vedendo quali erano i risultati della della riforma che era in corso; no, la fretta elettorale fa sì che la vostra scadenza sia il 26 maggio, in cui si parlerà di altro (sono le elezioni europee). Per voi, per la vostra sopravvivenza e per una parte di coalizione del Governo,

Presidente, rappresentanti del Governo, care colleghe e cari colleghi, l'Italia è un Paese bellissimo, è una terra bellissima per la composizione morfologica dei suoi territori, suoi territori, ma anche perché l'ingegno e lo spirito di iniziativa e di intrapresa degli italiani hanno sempre rappresentato il grande valore aggiunto della nostra Nazione, rendendola unica. L'Italia è sempre stata anche un Paese estremamente solidale e attento alla salvaguardia e al sostegno delle fasce più deboli, a tutti i livelli (economico, sociale e sanitario) e ha un sistema del *welfare* organizzato e capillare a livello locale, regionale e nazionale. l'Italia, proprio per la naturale e secolare vocazione al lavoro, all'intrapresa, all'artigianato, alla creatività, alla ricerca, alla crescita culturale e scientifica, culturale e scientifica, non è mai stata un Paese che si sia accontentato di iniziative di puro assistenzialismo, che annichiliscono queste attitudini, soprattutto nei giovani, minandone la dignità. Questo è delittuoso. Quello che approda oggi nell'Assemblea del Senato è il provvedimento più identitario di questo Governo: contiene le due misure che hanno condizionato la trattativa con la Commissione europea e che hanno determinato un *iter* di approvazione, vogliamo dire, anomalo (per non dire altro) della legge di bilancio; anomalo e ai limiti della correttezza formale, per chi ha ancora il senso delle istituzioni che rappresentiamo. Pertanto, per come è strutturato, noi non possiamo sostenere questo provvedimento. Noi non lo possiamo sostenere soprattutto nella parte che riguarda l'attribuzione di un reddito di cittadinanza che, nel tentativo goffo e inefficace di combinare il sostegno alla povertà e l'avviamento al lavoro, è invece destinato a trasformarsi in una misura puramente assistenzialista, un'inutile, umiliante, dannosa elemosina, priva di ogni effetto benefico sulla produttività e sui consumi e disincentivante per la ricerca di lavoro; misura peraltro destinata a pochi (circa 1,3 milioni su 5 milioni) e probabilmente nemmeno i più bisognosi, che determina un massacro burocratico e un utilizzo del debito che creerà un buco difficilmente colmabile. Tutti Tutti riconosciamo e vogliamo sostenere il bisogno, ma che lo si preveda come posta di crescita è pazzesco, perché in questo modo si può solo disincentivarla. Noi la nostra ricetta l'abbiamo rivelata attraverso gli emendamenti. Si chiama quoziente familiare, si chiama *flat tax* vera, si chiama riduzione del cuneo fiscale, si chiama defiscalizzazione per sei anni per le nuove assunzioni. Tutto procede, tra l'altro, tra confusione e pasticci, tanto che nulla è pronto per prendere in carico il beneficiario al momento, che arriverà, dell'erogazione del reddito previsto per il primo di aprile, nelle piattaforme, nei centri per l'impiego, nei CAF, nei Comuni o nelle Regioni. Non parliamo dei Comuni e delle Regioni, enti che saranno messi in seria difficoltà perché sulle loro spalle, come al solito, ricadrà molto del peso economico e organizzativo. Sono ben lontane le assunzioni dei quattromila addetti previsti nella legge di bilancio per i centri per l'impiego, così come i contratti di collaborazione per i 6.000 *navigator* presso ANPAL Servizi. E qui si crea un paradosso perché, mentre il Governo dice di voler cancellare il precariato, con questo provvedimento crea altri precari, precari di Stato. Oggi, infatti, siamo chiamati a votare un provvedimento per il quale le risorse sono state stanziate fino al 2021. E poi, che fine faranno questi lavoratori? Senza il lavoro, che non si crea dal nulla, ma sostenendo i datori di lavoro e formando al meglio i futuri lavoratori rispetto alla domanda, senza il lavoro si creeranno cittadini dipendenti dal reddito di cittadinanza, con la conseguenza che, quando questo reddito verrà rimosso, perché verrà rimosso, gioco forza, quel milione e passa di persone che hanno rinunciato al lavoro e alla formazione naturale si troveranno inoccupabili, cioè senza capacità e metodo per inserirsi nel mercato del lavoro. *(Applausi dal una droga illusoria, che crea dipendenza e distrugge la libera iniziativa soprattutto nei giovani, lasciandoli annichiliti. Ripeto che questo è delittuoso. Ci vuole ben altro per creare posti di lavoro. Bisogna attivarsi per diminuire, da un lato, le tasse e, dall'altro, la burocrazia; per intervenire, come dicevamo, sul cuneo fiscale e creare infrastrutture, FI-BP)*. Bisogna rendere competitive le nostre imprese con quelle straniere, attivare accordi con i Paesi stranieri per incrementare l'*export.* Solo così si crea lavoro, non solo con piccoli sgravi contributivi, oltretutto a rischio penale. Non si può e non si deve agire al ribasso, al livellamento verso il È necessario, invece, mettere in campo misure che stimolino la crescita, non solo economica e lavorativa, ma anche personale, soprattutto nei giovani. Divano e lavoro nero non possono essere gli obiettivi di un Paese come l'Italia, il Paese dell'Umanesimo, il Paese del Rinascimento, il Paese di Leonardo Da Vinci. Quota 100: la riforma del sistema pensionistico era ben presente nel programma con cui il centrodestra si è presentato alle scorse elezioni politiche, ma non lo era certo al ribasso, come, invece, sembra essere stato affrontato in questo provvedimento. Capisco, però, che così Innanzitutto, va rilevata la stranezza per la quale le disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno sessantadue anni di età e trentotto anni di contributi siano solo in via sperimentale e per il triennio 2019-2021. Quindi, è un provvedimento limitato nel tempo e che, in ogni caso, avvantaggia un numero altrettanto limitato di persone. Ora, posto che sia ragionevole e di buon senso garantire la flessibilità in uscita a chi vuole andare in pensione prima, non possiamo non evidenziare come questa sia una riforma molto costosa, a danno delle giovani generazioni che si troveranno a pagare un'altra ipoteca sul futuro dei nostri figli. La flessibilità in uscita dal mondo del lavoro attraverso le pensioni andrebbe contemperata da un maggiore ingresso nel mercato del lavoro. Ed è evidente come questo cozzi con la misura assistenzialistica del reddito di cittadinanza. A quota 100, in previsione, aderiranno 320.000 lavoratori, 200.000 del comparto privato e circa 100.000 del pubblico, all'interno, però, di categorie importantissime: medici, insegnanti, pubblica amministrazione, l'INPS per prima, creando un vuoto nel *turn over* nel pubblico e non necessariamente, invece, creando nuove assunzioni In conclusione, possiamo dire una sola cosa. Questo provvedimento è un provvedimento bandiera, bandierina. Serve esclusivamente a far credere agli elettori, prima delle elezioni europee, di aver mantenuto le promesse della campagna elettorale. elettorale. È giusto ricordare, ancora una volta, che per riuscire a portare a casa entrambe le misure di questo decreto-legge siete dovuti ricorrere al *deficit*. Tutto perché nessuno dei due partiti di Governo ha accettato di cedere sul proprio cavallo di battaglia, almeno a livello di tempo e di priorità. Come si può anche solo pensare di unire una misura di assistenzialismo e di diseducazione al lavoro come il reddito di cittadinanza con delle misure di avviamento al lavoro, utili e, anzi, necessarie per sostenere gli esiti di quota 100, che svuoterà di fatto solo alcuni comparti? Sarebbe bastato poco. La questione per noi è trovare le giuste soluzioni e dire no alla crescita infelice. Questo Paese non ha bisogno di stampelle per tenersi in piedi, come fa, invece, questo Governo che per restare in piedi crea decreti *ad hoc* per non scontentare tutti, ma senza accontentare nessuno. non ha bisogno di stampelle perché non può e non deve restare solo in equilibrio; ha bisogno di scarpe nuove e di piste veloci su cui correre. Basta bugie! Il lavoro è l'unica forma possibile di contrasto alla povertà.

il reddito di cittadinanza è evidentemente molte cose. È una misura contro la povertà, per l'accompagnamento al lavoro e per l'emersione del nero. È molte cose; lo abbiamo già sentito in parte degli interventi dei colleghi e sono certa che molto ancora potremo udire nella discussione che seguirà. Oggi mi piacerebbe soffermarmi sull'enorme potenziale di trasformazione culturale che questa misura porta con sé. con sé. Il reddito ha in verità molto a che fare con la nostra volontà di decidere se riconoscerci uguali sul piano esistenziale e avviarci a una decisa evoluzione culturale o diversi per diritto di nascita e abdicare per sempre all'attuazione della nostra Carta costituzionale. Ho la convinzione che il fondamento di ogni ingiustizia risieda nell'idea, molto umana purtroppo tra le idee umane, che tutti Grazie Si diventa, perciò, innocenti e inerti rispetto al dolore del mondo perché se nasciamo con diritti diversi legittimi diventano i destini diversi. Questa è purtroppo un'idea evidentemente presente anche nella nostra sottocultura, nel disegno di tutte le prime e seconde classi dei nostri percorsi di vita, perché è una componente latente di tutti i Paesi fatti È un'idea che appartiene a tutte le società fatte

è una nostra zavorra culturale perché, dove non è più il lavoro, lo studio e l'applicazione alla personale eccellenza di ciascuno il motore della promozione sociale, ma la sola capacità di guadagnarsi l'accesso alle linee di potere, i parametri tribali delle differenze sacrali tra gli uomini si sostituiscono sempre a quelli razionali dei diritti equi. Oggi a noi italiani piace distinguerci gli uni dagli altri, ma perché non ci è stato lasciato molto altro, oltre la distanza che mettiamo gli uni verso gli altri, per consentirci di innalzare noi stessi. Questa componente culturale - che chiamerei «il piacere delle differenze» - si porta dietro, purtroppo, come suo logico compagno il disprezzo per l'altrui caduta sociale e come suo naturale corollario la disoccupazione indicata come colpa evidente e la povertà come destino meritato. Ma quanto è colpevole colui che non trova lavoro in un Paese in cui nessuno mai si è preoccupato di rendere evidente il lavoro? In quanta parte è responsabile per il suo destino un uomo inginocchiato nella depressione e nella rassegnazione all'interno di un sistema economico-produttivo dichiaratamente e matematicamente costruito a ingresso limitato? Ai nostri provincialismi si aggiunge poi una difficoltà oggettiva: che sia difficile e quasi innaturale per coloro che fortunatamente continuano a godere di protezione e benessere, in una società in cui povertà e disoccupazione crescono esponenzialmente, riuscire a figurarsi l'ombra infinita che intanto attraversa in quella stessa società chi è senza mezzi e senza lavoro; l'infinita sequela di umiliazioni e la conseguente discesa interiore fino alla certezza, in se stessi per primi, di essere indegni di benessere e meritevoli di fallimento. Perciò non era facile arrivare al reddito di cittadinanza in Italia. Il valore attribuito alla distanza sociale, la colpa ascritta alle fragilità, l'impossibile empatia delle minoranze economicamente avvantaggiate hanno lungamente sbarrato il passo alla civiltà profonda insita in questa riforma. Non era per niente facile, perciò oggi io non posso nascondere l'orgoglio di far parte di una forza politica che ha saputo guardare oltre tutte le nostre piccolezze, i nostri immobilismi e immaginare e volere per noi un destino infinitamente più grande

diffusa. Quando avremo sollevato lo sguardo dalle nostre piccole guerre col vicino non resterà altro da fare in campo che guardare avanti e rivolgersi all'idea di diventare grandi e questo è un destino per la nostra Nazione che tutte

che soprattutto rispondesse a una esigenza di giustizia che ci chiedevano i cittadini. Noi abbiamo assunto questa esigenza come impegno e per essa abbiamo combattuto negli ultimi cinque anni, da quando è stata varata una riforma che ha modificato il sistema pensionistico italiano, trasformando un modello che, partito negli anni Ottanta dalle *baby* pensioni, è arrivato a prevedere un'età pensionabile fra le più alte in Europa. È evidente che

rispetto alla quale non c'è stata una manifestazione di protesta significativa da parte mondo sindacale, che oggi protesta non si sa bene per quali riforme varate da questo Governo. Ricordo invece che quella riforma è stata votata dalle stesse forze politiche che oggi criticano questo nostro provvedimento, che non sarà perfetto ma va nella direzione giusta Questo è semplicemente un atto di giustizia. C'è chi ritiene che non sia adeguato e sufficiente, eppure chi critica il provvedimento in questi termini cinque anni fa ha votato

Noi invece riteniamo che di fronte a un sistema pensionistico ingiusto, in occasioni come queste non ci si debba porre tante domande, ma solo chiedersi se è giusto modificare questo sistema. Per noi

Noi non rendiamo giustizia esclusivamente a coloro a cui è negato il diritto di andare in pensione a un'età dignitosa. Noi rendiamo giustizia anche alle nuove generazioni che ancora in quest'anno e negli anni passati sono state costrette a lasciare il nostro Paese, ad abbandonare l'Italia

di entrare nel mondo del lavoro ai nostri giovani o a coloro che, meno giovani, ne sono stati espulsi: è una grande opportunità che va colta. Abbiamo assunto questo impegno sin dall'inizio, abbiamo fatto la campagna referendaria e abbiamo raccolto più di 500.000 firme per cambiare questa legge. Solo la Corte costituzionale ci ha impedito che si tenesse quel *referendum*, ma i cittadini hanno capito che potevano riporre fiducia nella Lega e ci hanno dato consenso il 4 marzo anche per questa battaglia. Siamo orgogliosi che, a meno di un anno da quelle elezioni, siamo in grado di presentare un provvedimento che non sarà perfetto, non renderà giustizia a tutti i lavoratori, ma è sicuramente un passo in avanti. Lo consideriamo un punto di partenza e non un punto d'arrivo.

ed è giusto tentare di dare una risposta anche a quelle famiglie che non hanno alcuna prospettiva, con l'impegno però che questo provvedimento - come abbiamo cercato di fare con la nostra azione emendativa porti a nuova occupazione. Questo è il nostro intendimento, è quanto abbiamo cercato di fare attraverso gli interventi dei nostri componenti in Commissione e sarà il ruolo che giocherà la Lega nell'attuazione di questa riforma.

reddito di inclusione. C'è dell'ipocrisia anche da parte degli amici alleati di Forza Italia, perché vorrei ricordare che in campagna elettorale qualcuno promise il reddito di dignità: 1.000 euro al mese garantiti per tutti. Questa persona è il *leader* di Forza Italia: lo era prima del 4 marzo e lo è anche oggi. Disse, in quella campagna elettorale, che chi è sotto una certa soglia di reddito non deve pagare le tasse,

in una fase concitata della campagna elettorale, ha cercato di introdurre tematiche che sicuramente non appartenevano alla nostra coalizione, ma sono state probabilmente introdotte alla ricerca di un consenso che veniva meno. Noi siamo orgogliosi di portare a compimento un impegno che abbiamo preso con gli elettori: il superamento della legge Fornero. È un impegno che avevamo preso e con determinazione e coerenza stiamo portando a compimento. Ripeto: è una partenza, ma possiamo dire con orgoglio che quella riforma non l'abbiamo votata e chi oggi ci critica sono le forze politiche che l'hanno varata e hanno avuto

votiamo questo provvedimento con convinzione, sicuri che porterà anche a maggiore occupazione per il nostro Paese, che è la vera priorità per gli italiani. *(Applausi

rivoluzione per il mondo del lavoro. L'opposizione cerca di sminuire la portata di questa legge, tutta l'opposizione, da destra a sinistra ovviamente. Il motivo è chiaro: cercano di nascondere la storia economica del nostro Paese degli ultimi trent'anni dietro a un muro di omertà, di approssimazione, di paura, di pessimismo, di mera strumentalizzazione politica, pensando di ingannare gli italiani. Loro possono provare a nascondersi, ma non possono nascondere i milioni di cittadini che, a causa della loro incapacità, sono entrati nel dramma della povertà, di una vita senza lavoro, di una mancanza di futuro per loro stessi e per la loro famiglia. A chiacchiere hanno sbandierato per anni il famoso articolo 1 della Costituzione; poi, come al solito, con le loro azioni politiche ne hanno fatto carta straccia. Le vittime di questa opposizione disconnessa dalla realtà, lontana anni luce dai reali bisogni dei cittadini e che per decenni ha governato il Paese non sono stati solo i cittadini più poveri e fragili, ma anche le classi medie, quelle che da sempre sono state la forza silenziosa e operosa che ha permesso all'Italia di diventare un Paese avanzato dal punto di vista economico e sociale. Troppo spesso le misure scellerate degli ultimi Governi si sono orientate a favore dei soliti portatori di interessi torbidi. Questa misura invece vuole riportare al centro il cittadino, sia quello più fragile (con misure concrete come il reddito di cittadinanza), sia quello appartenente alla classe media, ormai entrata nel limbo di una vita priva di lavoro, di prospettive e di speranza per il futuro loro e dei loro figli. Noi questa speranza e questa prospettiva vogliamo restituirla loro. Abbiamo preso l'impegno con i cittadini e lo stiamo mantenendo: nessuno deve rimanere indietro e nessuno rimarrà indietro. Le misure di questa legge, infatti, sono chiare, concrete e vanno a toccare i punti deboli del sistema del lavoro, con massicci interventi di politica attiva. Nei centri per l'impiego di Germania e Francia, per esempio, lavorano rispettivamente 100.000 e 54.000 addetti; in Italia sono 8.000.

Nessuno; ma questo Governo, il Governo di cui fa parte il MoVimento 5 Stelle, sì. La riforma dei centri per l'impiego, che costituisce una vera e propria riforma strutturale del mercato del lavoro, ha come obiettivo quello di rimettere in gioco

i centri per l'impiego permetterà di rivedere al rialzo il tasso di partecipazione alla forza lavoro, con conseguente crescita anche del PIL potenziale. I centri per l'impiego rappresentano il fulcro del sistema pubblico per dare lavoro a giovani e meno giovani; e abbiamo incontrato persone estremamente preparate nei centri per l'impiego. Questi centri per l'impiego, così bistrattati da chi li ha gestiti male per decenni, oggi noi vogliamo rimetterli al centro, potenziandone capacità e professionalità. Mentre per anni i centri per l'impiego sono stati trascurati, depotenziati, snaturati nella loro importante funzione sociale, noi

La riforma dei centri per l'impiego, che costituisce una vera e propria riforma strutturale del mercato del lavoro, ha come obiettivo quello di rimettere in gioco oltre 3 milioni di scoraggiati, che da anni nemmeno provano più a cercare attivamente un lavoro. L'afflusso di questi scoraggiati presso i centri per l'impiego permetterà di rivedere al rialzo il tasso di partecipazione alla forza lavoro, con conseguente crescita anche del PIL potenziale. I centri per l'impiego rappresentano

noi oggi abbiamo trovato i mezzi economici e la convinta volontà politica di fornire loro rinnovata forza propulsiva, mettendo di nuovo a fianco del cittadino in cerca di lavoro questi uffici determinanti per le origini del lavoro. Poi, sempre in tema di politiche attive e di reinserimento nel mercato del lavoro, possiamo citare sia l'articolo 8, che prevede incentivi per le imprese che assumono il beneficiario del reddito cittadinanza a tempo pieno pieno e indeterminato, sia l'articolo 9 che prevede, quale strumento di inserimento lavorativo, l'assegno di ricollocazione. Si tratta, in concreto, di una somma di denaro che il lavoratore potrà spendere presso enti accreditati dai centri per l'impiego che gli permetterà di ricevere un servizio di assistenza intensiva per la ricerca di occupazione con la finalità di aiutare la persona disoccupata a migliorare la possibilità di ricollocarsi nel mondo del lavoro, configurandosi quindi come una concreta misura di politica attiva. Per concludere mi rivolgo alle opposizioni, da sinistra a destra: ci avete consegnato un Paese con cinque milioni di poveri, l'abbiamo detto in molti. Soltanto pochi anni fa erano un milione e mezzo. Avete minato la vita delle classi medie e trovate anche il coraggio di criticare la nostra riforma. In questi giorni vi abbiamo sentito protestare perché, secondo voi, il reddito di cittadinanza è di importo troppo elevato. Veramente il vostro obiettivo politico, la vostra ambizione è quella di togliere 30, 40 o 50 euro ai cittadini italiani in difficoltà? Il vostro è un atteggiamento che si commenta da solo. Mi permetto un consiglio: fermatevi, pensate e riflettete. Potrete cercare di propinare i soliti vecchi discorsi, le solite parole vuote, le ormai famigerate *fake news*, ma la realtà è limpida e oggettiva e la vogliamo ribadire ad alta voce con poche, chiare parole: questa è una riforma per tutti, per restituire dignità a milioni di persone e per ridare un futuro all'Italia.

Signor Presidente, alcuni interventi dei colleghi della maggioranza mi stavano spingendo a stracciare il mio intervento e provare a recitare magari «I Miserabili» di Victor Hugo, Steinbeck, magari discettare sulla «Laudato si'» di papa Francesco o sulla dottrina sociale della Chiesa, perché mi pareva che il tono fosse questo, la riflessione fosse di questo tenore. ci sto volentieri anche a parlare della globalizzazione, della carità, del Vangelo. Però stiamo parlando oggi di questo decreto-legge e - ahimè - mi tocca tornare coi piedi per terra, nella vita, perché qui al Senato non stiamo parlando di Victor Hugo, di Gramsci (grandissimo)

e non sui massimi sistemi, su cui possiamo discettare e credo potremmo dedicare una serata intera sui problemi della crisi dell'Umanesimo e di tutto quello che si vuole. E allora provo, Presidente, a tornare nel merito del provvedimento. Si può essere contro un provvedimento che si pone l'obiettivo di contrastare la povertà? Ovviamente no, a patto che il provvedimento vada nella direzione giusta e che si faccia bene il bene. Si faccia bene il bene. al nostro esame il bene che proponete - lo dico con molto rispetto della maggioranza - è confuso e intriso di una burocrazia asfissiante. Basta leggere il testo: è una sequenza di procedure e di tempistiche irrealizzabili, una paranoia di efficienza che nulla ha a che vedere con l'efficienza che attiva il bene. E a pagare saranno i poveri. Il ministro Di Maio soltanto alcuni mesi fa dichiarava che sarebbe stata cancellata la povertà. Una dichiarazione impegnativa, ma non sarà così. Ahimè, non saranno coinvolti tutti i 5 milioni di poveri assoluti nel Paese. Saranno probabilmente soltanto 3 milioni e un quarto di quella platea che viene in qualche modo censita dall'Istat, sarà esclusa. Non sono dati del Partito Democratico, ma sono i dati che abbiamo ascoltato che abbiamo ascoltato tutti, come può testimoniare la presidente Catalfo, dai sindacati, dall'Ufficio parlamentare di bilancio, da Confindustria, da Alleanza contro la povertà, dalla Caritas, dalla Conferenza episcopale italiana. Sono dati che riportiamo semplicemente come annotazioni critiche che dovrebbero essere ascoltate.

quindi un diritto per tutti. È un diritto a tempo determinato. Spiace dirlo al vice presidente Di Maio; è a tempo determinato perché se le risorse non saranno sufficienti, il diritto verrà rimosso. Altro che rivoluzione del *welfare*, cambiamento e misure universalistiche. State creando un'aspettativa che produrrà ancora più delusione ed incertezza. Le persone e le famiglie fragili tanto evocate nei vostri interventi non meritano illusioni e false speranze.

Victor Hugo, la «Divina commedia» e i «Promessi sposi». La prima di queste osservazioni è che il provvedimento confonde due linee di *policy* che l'esperienza insegna a tenere ben distinte: quella del contrasto alla povertà e quella delle politiche attive del lavoro. Può infatti accadere, cari colleghi, che un povero non sia occupabile per motivi suoi, di vita, e può accadere che un disoccupato non sia in condizioni di povertà e che abbia bisogno di formazione, di una ricollocazione nel sistema produttivo del territorio.

di sinistra o comunisti - che soltanto il 20 per cento dei beneficiari sono ricollocabili. Gli altri non lo sono. Lasciate senza protezione i disoccupati. Quindi non tenete conto dei poveri e dei più poveri e lasciate senza protezioni i disoccupati. Povertà sociale e povertà di reddito vanno distinte: la povertà di reddito si combatte con l'occupazione, producendo lavoro, mentre la povertà sociale si combatte con la presa in carico. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Sono due percorsi diversi: abbiate pazienza, colleghi, ogni tanto ascoltate! La ogni tanto ascoltate! La povertà sociale ha bisogno di presa in carico, di attenzione, di una collaborazione del territorio e della comunità. La povertà di reddito ha bisogno di investimenti e coloro che possono produrre investimenti e lavoro sono le imprese, che in questo testo neppure avete citato, semmai incaricandole e appesantendole di altre incombenze.

che hanno la sola colpa di essere famiglie straniere, pur regolari. Si colpiscono le 30.000 persone senza fissa dimora, i più poveri tra i poveri. Si chiedono verifiche patrimoniali improbabili alle famiglie straniere, che avete introdotto per giustificare e dare una copertura normativa a quanto è accaduto a Lodi. È una tristezza infinita, altro che diritti! Si colpiscono persino gli italiani residenti all'estero, che tornando a casa, in Italia, in caso di bisogno non potranno accedere ad alcun beneficio. È questa la cosa che sta accadendo, sono questi i dati di realtà, perché la politica è fatta di realtà e non di sogni filosofici. Si tratta dunque di provvedimenti che ledono i diritti costituzionali, perché per noi vengono prima le persone, tutte le persone, senza se e senza ma,

irrealizzabili. La prima fragilità sono i centri per l'impiego: avevate promesso durante la campagna elettorale che avremmo atteso una grande riforma dei centri per l'impiego prima di introdurre il reddito cittadinanza. Lo avete detto e invece avete improntato un impianto

inclusione avevamo proposto un percorso diverso, perché un pochino la povertà l'avevamo studiata. Ci abbiamo messo non perché il provvedimento fosse così complicato, ma perché un provvedimento di questo tipo lo si fa ascoltando la realtà e la vita. Bisogna conoscere le cose: i poveri bisogna un po' conoscerli e non si può soltanto declamare sulla povertà.

potenziare quell'esperienza. Avete però rinnegato tutto, facendo perdere tempo al Paese un'altra volta e credendo che il cambiamento avvenga sul nulla. Il cambiamento, quello buono e proficuo, avviene quando si innestano azioni positive su quanto di buono è stato fatto. Il Rei aveva

per contrastare la povertà. Voi di questo non avete parlato, addirittura avete appesantito i Comuni di altri impegni burocratici, li avete praticamente resi resi inetti, impossibilitati ad agire in questo senso. Questa è la vostra riforma, una riforma che non darà speranza, una riforma che creerà più povertà, in un momento difficile che sta attraversando il Paese. Voi farete una manovra di nove, dieci miliardi (Tria dice che non si farà, ma Tria è una persona seria e immagino che la si farà). Quindi, con questo provvedimento date dieci miliardi e fra qualche mese

oggi è davvero un bel giorno per essere del MoVimento 5 Stelle, perché abbiamo l'occasione di realizzare il nostro sogno di migliorare la qualità della vita di tanti italiani e al contempo di mantenere fede agli impegni che abbiamo preso in campagna elettorale. Finalmente stiamo per approvare in quest'Aula un provvedimento che racchiude in sé quattro capisaldi della nostra proposta politica: la lotta alla povertà e il miglioramento delle politiche attive per il lavoro che conseguiamo per mezzo del reddito di cittadinanza, l'innalzamento delle pensioni mediante la pensione di cittadinanza e infine il superamento della famigerata legge Fornero, con la cosiddetta quota 100. Il cammino per arrivare in quest'Aula è stato lungo, difficile e tortuoso. Noi ci abbiamo sempre creduto, anche quando i soloni della politica e i grandi commentatori dei giornali ci dicevano che non ci saremmo mai riusciti, che appena arrivati al Governo avremmo cambiato idea e che l'Europa non ce l'avrebbe permesso, che avremmo dimenticato le promesse elettorali come fanno tutti gli altri. *(Applausi invece no, siamo qui al servizio dei cittadini, al servizio di chi in questo momento soffre e ha bisogno di aiuto da parte della collettività e si affida con fiducia allo Stato, lo Stato che deve essere solidale ed equo, non piegato agli interessi di pochi e agli interessi delle *lobby*. I detrattori in servizio permanente effettivo ci accusano di approvare il reddito di cittadinanza in questo momento per una mera convenienza elettorale, voglio ricordare loro che è passato già un anno dalle elezioni: quanto altro tempo ancora i nostri connazionali devono soffrire, quanto devono aspettare, chi lo stabilisce quando dobbiamo approvare questo provvedimento? Del resto, se lo avessimo fatto, come voi ci consigliate, l'anno prossimo, ci avreste detto che lo facevamo perché era in funzione delle elezioni regionali e così via, e quindi si sarebbe perpetuato questo discorso. Noi invece siamo fieri di approvare questo provvedimento dopo solo otto mesi

a dismisura in pochissimi anni a causa delle folli politiche di austerità imposte dall'Europa e abbracciate dai Governi italiani: Monti, Letta, Renzi, Gentiloni Silveri. Voi avete fatto queste politiche. Il reddito di cittadinanza cambierà radicalmente la situazione, perché non sarà solo un sussidio, ma verrà affiancato da un sistema efficiente e articolato di politiche attive del lavoro, incentrato sui centri per l'impiego. è prevista l'assunzione di 4.000 nuovi operatori qualificati, che si aggiungeranno agli attuali 8.000 (che sono davvero pochini, se li confrontiamo con quelli di Francia e Germania, come ha detto poc'anzi il collega Romagnoli); altri 6.000 saranno assunti da ANPAL come *navigator*, che prenderanno in carico i beneficiari del reddito di cittadinanza per accompagnarli passo passo verso un nuovo impiego. Per diventare *navigator* occorrerà avere una formazione, quindi una laurea magistrale in economia, giurisprudenza, sociologia, scienze politiche, psicologia o scienze della formazione. Inoltre, altro aspetto molto importante, si realizzerà il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che sarà collegato al sistema informativo unitario dei servizi sociali, il che permetterà di interconnettere tutte le banche dati esistenti, in modo tale che si conoscano formazione e competenze di ogni lavoratore, sì da incrociarle con le esigenze e le richieste delle aziende presenti su tutto il territorio nazionale. L'investimento complessivo nelle politiche attive del lavoro sarà di 2 miliardi nel biennio 2019-2020. Questi investimenti aiuteranno a colmare il *gap* che in questo settore esiste tra il nostro Paese e tutti gli altri Paesi europei e che è figlio delle politiche miopi dei Governi precedenti, che non hanno mai preso seriamente la questione delle politiche attive del lavoro. in campagna elettorale avevamo promesso di superare la famigerata legge Fornero, istituendo quota 100, favorendo il ricambio generazionale, liberando posti di lavoro per i giovani, rinnovando e migliorando le competenze della forza lavoro e quindi, in definitiva, avviando a soluzione quel conflitto generazionale che ha costretto centinaia di migliaia di ultrasessacinquenni a rimanere sul posto di lavoro e, nel contempo, altrettanti giovani alla disoccupazione o all'emigrazione.

versati e inoltre, se si sono maturati questi requisiti entro il 2018, si potrà andare in pensione già dal 1º aprile 2019; se invece si matureranno nel corso del 2019, si potrà andare in pensione

Tutti i dipendenti pubblici, sia coloro che sceglieranno quota 100, sia gli altri, riceveranno da subito la prima rata del TFR o dell'equivalente fino a 45.000 euro. Un'altra importante novità è che gli iscritti a due o più gestioni previdenziali che non siano titolari di pensione potranno cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stessi gestioni amministrate dall'INPS per accedere a quota 100. inoltre abbassato i requisiti per accedere alla pensione anticipata e quindi, dagli attuali quarantatre anni e cinque mesi di contributi per gli uomini, si scende a quarantadue anni e dieci mesi, cioè sette mesi in meno, mentre per le donne il risparmio è di un anno, a prescindere dall'età anagrafica. Ebbene, noi amiamo questo nostro Paese e siamo oggi emozionati e felici, perché sta per concludersi la prima tappa di un lungo cammino iniziato dai nostri fondatori Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio *(Applausi dal Gruppo e noi la stiamo percorrendo insieme ai cittadini che hanno creduto nel MoVimento 5 Stelle e ci hanno votato. *(Applausi

Ma l'hanno studiata, ed è già qualcosa. Per comprendere l'importanza del provvedimento che stiamo discutendo oggi e che ci apprestiamo a votare in quest'Aula, della sua portata e degli effetti benefici che avrà sul popolo italiano, nel mio intervento mi sia concesso di prendere in prestito, quasi come un tributo, alcune celebri parole pronunciate da Roy Batty. Perché in merito alle pensioni, alle riforme promosse negli scorsi anni e al dibattito che è stato portato avanti dalle diverse forze politiche al riguardo, ci sarebbe tanto da dire. E dunque potrei affermare che, sotto questo aspetto: «io ne ho viste di cose che voi umani non potreste immaginarvi». e M5S).* Signor Presidente, ho visto un Governo legittimo che, sostenuto da una maggioranza parlamentare eletta dal voto dei cittadini, è stato costretto alle dimissioni, portato a esaurire il proprio mandato sulla base di ordini dall'alto, di pressioni da parte delle *lobby* e delle alte finanze internazionali, a colpi di *spread*, con buona pace del risultato delle libere elezioni con cui il popolo italiano si era liberamente espresso. Ho visto arrivare subito dopo un nuovo Governo che per nulla rappresentava i cittadini, piazzato lì per volere degli stessi che avevano spinto per la caduta di quello prima, frutto di una manovra di palazzo. Il Governo dei professori, dei *loden*, di quelli che dovevano salvare l'Italia, ma che invece hanno fatto l'esatto opposto, mettendo gli interessi dell'Italia e degli italiani all'ultimo posto della loro agenda amministrativa. Per anni abbiamo dovuto ingoiare le loro pessime riforme e le loro scelte sbagliate, sempre accompagnate dal bollino «ce lo chiede l'Europa». Mai una volta che avessero detto: «Ce lo chiedono gli italiani». Ho visto Ministri piangere per le loro stesse riforme. La legge Fornero, ce la ricordiamo tutti, purtroppo. Ce la ricordiamo noi, che l'abbiamo combattuta, e nessuno se lo dimentichi. Se la ricordano i giovani, gli esodati, i lavoratori che hanno dovuto subirla. Un provvedimento iniquo che grida vendetta, votato nel 2011 in Parlamento dalla coalizione di partiti che sosteneva il Governo Monti: PD, PdL, Unione di Centro, Futuro e Libertà per l'Italia e altri Gruppi. La Lega votò contro, sempre coerenti e contrari a una legge ingiusta, che andava abolita. Matteo Salvini e la Lega l'avevano promesso e lo stiamo facendo, passo dopo passo: ancora una volta dalle parole ai fatti. Ho visto associazioni, intellettuali, sindacati sempre pronti a lanciare accuse contro questo Governo o a scendere in piazza per manifestare il proprio dissenso, che poco o nulla hanno fatto per osteggiare o bloccare la legge Fornero, dando così ragione a chi sostiene che molto spesso certe sigle sono più preoccupate di difendere la propria esistenza o le proprie posizioni di potere, anziché difendere realmente i diritti dei lavoratori e in particolare degli italiani. Ho visto partiti politici che sono stati capaci di sostenere senza alcuna vergogna i Governi Monti e Letta, e di dare il proprio sostegno ai provvedimenti portati avanti da questi Governi, che hanno certamente e indiscutibilmente portato l'Italia sull'orlo del baratro e impoverito le famiglie, i lavoratori, i pensionati e quindi gli italiani. Per poi, oggi, pochi anni più tardi rispetto all'approvazione di quella vergognosa riforma, indossare i *gilet* blu contro questo Governo che sta tentando di porvi rimedio. Io mi vergognerei. Gentile Presidente, come dicevo poc'anzi, ho voluto omaggiare Roy Batty per elencare le assurdità, le storture e le scelte sbagliate di chi ci ha preceduto. Nemmeno in «Blade runner», meraviglioso film di Ridley Scott, si sono viste cose così incredibili. Anche se non sono il grande attore Rutger Hauer, faccio mia la frase recitata nell'ultima epica scena. Lui diceva che «tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia». Ebbene questo non è il nostro caso, perché nessuno di noi dimentica quanto successo negli ultimi anni; grazie a Matteo Salvini, alla Lega e a questo Governo siamo qui per cambiare le cose. Il contratto di Governo lo dice chiaro: occorre prevedere l'abolizione degli squilibri del sistema previdenziale introdotti dalla riforma delle pensioni

lo abbiamo promesso, lo facciamo e lo faremo. Perché questo non è un punto di arrivo, si badi bene, ma un punto di partenza per smontare la legge Fornero e superarla, dando risposte concrete ai cittadini, dando la speranza di un futuro ai nostri ragazzi, consentendo a chi ha lavorato tutta la vita di godersi finalmente la meritata pensione. Siamo convinti che, laddove si ripristina la libertà di scegliere se andare o meno in pensione, si regala dignità agli uomini e alle donne che hanno lavorato per tutta la vita; si consente loro di scegliere, signor Presidente. Sì, di scegliere; in un momento storico in cui tutto ci è imposto, questo Governo consente alle persone di scegliere il proprio futuro. Abbiamo solo ascoltato, abbiamo solo avuto la forza e l'umiltà di ascoltare il grido di coloro ai quali quella dignità era stata tolta; lo ha fatto Matteo Salvini, lo ha fatto questo Governo, lo stiamo facendo noi in quest'Aula. con il loro voto contribuiranno ad approvare questa riforma dico: siatene veramente orgogliosi e, quando ritornerete nei vostri territori, fatelo a testa alta, perché oggi è il giorno in cui gli italiani hanno vinto la loro partita, riprendendo finalmente in mano il loro futuro. È tempo di cambiare. Grazie Signor Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, il reddito di cittadinanza è un provvedimento che non creerà un solo posto di lavoro e sarà totalmente inutile e inefficace contro la povertà. Chi pensa che il reddito di cittadinanza possa dare una spinta all'occupazione dimostra di non conoscere né come funziona il sistema produttivo italiano, né, tanto meno, le regole del mondo del lavoro. La disoccupazione, cari colleghi, si combatte solo creando nuovi posti di lavoro e mettendo le aziende in condizione di assumere. Sarebbe stato, quindi, utile proporre politiche fiscali vere per chi assume. Infatti, per consentire che le attività e le aziende italiane siano in attivo e possano produrre reddito occorre fare poche cose ma diminuire le tasse e la burocrazia, incentivare l'economia aumentando gli investimenti nazionali e aprendo alle grandi opere pubbliche, esattamente il contrario di quello che sta facendo questo Governo.

prima date le offerte di lavoro e poi il reddito. Potenziate i centri per l'impiego con 4.000 assunzioni. Ricordo comunque al Governo che si devono ancora stabilizzare i 1.600 assunti un anno fa. Assumete 6.000 *navigator* per indirizzare le persone alla ricerca di un lavoro e questi saranno gli unici posti di lavoro che riuscirete a creare; saranno gli unici posti di lavoro che questo provvedimento creerà. Se, poi, è vero che si parla di una potenziale platea di 5 milioni di persone che potrebbero richiedere il reddito, significa - vorrei fare una riflessione insieme a voi - che ogni *navigator* dovrà occuparsi di circa 800 persone: una follia. Profili diversi, situazioni diverse, esigenze diverse, criticità diverse, gestiti da persone che non avranno un formazione adeguata in riferimento ai tempi di attuazione, così brevi, e che non sappiamo ancora come e da chi saranno assunti. La ricerca del lavoro verrà fatta da chi ora sta cercando un lavoro, ma che da marzo verrà chiamato *navigator*; in questo modo non funzionerà, perché per trovare perché per trovare un lavoro ad altri bisogna avere competenze tecniche e conoscenze del territorio e del sistema economico di riferimento. Ma poi tutto è concentrato - permettetemi - su chi chiede lavoro, e non c'è niente su come saranno acquisite le richieste di manodopera. Come faranno i centri per l'impiego a sapere qual è l'offerta di lavoro delle aziende? Quale strumento si metterà in campo per sapere di che tipo di manodopera e, soprattutto, quale azienda ne ha bisogno? Di tutto questo non c'è traccia nel testo. Molte realtà non si rivolgono ai centri per l'impiego. In agricoltura, ad esempio, solo il 2 per cento delle aziende si rivolge a questo tipo di centri per cercare manodopera. Bene, cosa volete fare per convincere l'altro 98 per cento? Noi non lo vediamo in questo provvedimento e forse neanche voi lo sapete. Ma almeno lo sapete quanto guadagna un bracciante agricolo stagionale? Guadagna tra gli 800 e i 900 euro al mese. E voi ne date 780 a chi sta comodamente a casa aspettando che qualcuno al suo posto si adoperi per cercargli lavoro. E se una persona ha l'obbligo di accettare l'offerta, vi siete posti il problema che l'azienda non ha l'obbligo di accettare chi gli verrà mandato? Se una persona non verrà accettata da nessuna azienda per la sua incapacità, cosa facciamo? Come ci si Come ci si dovrà comportare? In tutto questo, vengono dimenticati i giovani italiani disoccupati che, magari, non hanno i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza, ma hanno necessità di essere accompagnati al reinserimento lavorativo. Il problema della disoccupazione può essere risolto, oltre che con minor tasse e minor burocrazia per le aziende, iniziando da una politica integrata del sistema scuola-lavoro, con una politica apposita volta a formare figure professionali necessarie alle aziende: questa è la strada giusta. Invece, è stato proposto un testo inefficace, lacunoso, scritto in fretta (così da essere approvato prima delle elezioni europee) e che dà mance elettorali senza creare occupazione. Il reddito di cittadinanza è per noi una forma di assistenzialismo che aiuta immigrati e furbi, dimenticando i veri poveri, le famiglie numerose, gli invalidi, e i più deboli. In questo modo, gli unici che non verranno aiutati sono gli italiani onesti che hanno veramente bisogno. Fratelli d'Italia ha proposto decine di emendamenti per limitare i danni del reddito di cittadinanza e per migliorare quota 100. Abbiamo, però, trovato un muro di arroganza politica che non ha voluto nessun confronto concreto. Per questo siamo dispiaciuti: non perché non siano stati accettati i nostri emendamenti, ma per la nostra Nazione.

Politiche fallimentari, che hanno causato un aumento esponenziale della povertà nel nostro Paese; fino a ben cinque milioni di poveri. L'eccezionale aumento della povertà assoluta, dovuto al ridursi dei livelli occupazionali e a un sistema di ammortizzatori sociali fino adesso fallimentare, ha reso necessari l'introduzione di misure di sostegno al reddito e percorsi di inclusione lavorativa tramite il potenziamento delle politiche attive del lavoro. Nel biennio 2011-2013 si è registrato il picco più alto di povertà della storia d'Italia in tempo di pace, proprio nel periodo delle politiche di "*austerity*" tanto care al Governo Monti e all'Europa. Gli italiani in povertà assoluta sono passati, in appena due anni, da due milioni e mezzo circa nel 2011 a ben più di quattro milioni nel 2013. Un ulteriore aumento si è registrato poi nel biennio 2014 -2016, quando i poveri assoluti sono passati a quasi cinque Ricordo i Governi di quegli anni, che già poco fa un mio collega ricordava, che hanno la responsabilità di questi dati infausti: i Governi Monti, Letta, Renzi. Non manca il Governo Gentiloni Silveri a questo triste appello. Nel 2017, l'incidenza della povertà assoluta nel suo Governo sulla popolazione italiana è salita all'8,4 per cento. Questo è l'amaro lascito del Governo Gentiloni Più di cinque milioni di italiani che non possono permettersi di accedere ai beni primari e ai servizi essenziali, per uno *standard* di vita accettabile. Ancora una volta, a soffrire di più di questo andamento economico è il Sud, dove i dati sono in aumento, sia per le famiglie che per i singoli. Ma anche il Nord non se la passa bene, purtroppo. Una famiglia su due in stato di povertà vive in casa di affitto, in maggioranza nelle metropoli dell'Italia settentrionale. Mentre tra le famiglie che vivono in una casa di proprietà una su cinque paga un mutuo. Abbiamo pensato a tutto questo e lo abbiamo fatto bene prevedendo un contributo per le famiglie che hanno contratto un mutuo e anche per quelle che pagano un canone di locazione. Le politiche del Governo Renzi nel biennio 2014-2016 non hanno avuto alcun impatto positivo sulla crescita; hanno pensato solo di erogare il *bonus* di 80 euro, una misera mancia di cui hanno beneficiato ben 10 milioni di italiani e che è costata ben 10 miliardi di euro, a debito sul futuro dei nostri figli, senza sortire alcun effetto sui consumi. Inoltre, la misura di contrasto alla povertà del Governo Gentiloni Silveri, poc'anzi nominata, oltre a essere un provvedimento soltanto di natura assistenziale, è stata assolutamente insufficiente a soddisfare l'intera platea dei poveri assoluti. Il nostro provvedimento, invece, prevede un contributo di ben 780 euro per i *single* e fino a 1.330 euro per le famiglie numerose, mettendo sul piatto 7 miliardi di euro, già stanziati nella legge di bilancio 2019. Mi sia consentito un ultimo dato prima di chiudere. Dei destinatari del reddito di cittadinanza in età da lavoro, il 60 per ha come titolo di studio il diploma di scuola secondaria di primo grado, mentre il 13 per cento possiede la licenza elementare o addirittura nessun titolo. Sono uomini e donne del nostro Paese anche questi e i Governi passati se ne sono dimenticati, salvo pensare a come aiutare banche e banchieri. Sono uomini e donne che non sono mai stati presi in considerazione dalle leggi di bilancio e dai programmi economici dei Governi passati. donne difficilmente oggi troverebbero lavoro se non pensassimo a formare questi nostri concittadini con un percorso personalizzato di riqualificazione professionale e di completamento degli studi che il nostro patto prevede per l'inserimento nel mercato del lavoro. Finalmente questi cittadini avranno la possibilità di guardare avanti e cominciare a ricostruire il proprio futuro. Per tutelare i più deboli, però, abbiamo previsto delle sanzioni per chi se ne approfitta. Non c'è scampo per i disonesti. Il nostro provvedimento introduce meccanismi di controllo molto seri che non lasciano spazio a chi non vuole impegnarsi. Stiano pure tranquilli i nostri detrattori; abbiamo pensato proprio a tutto. Si preoccupino, invece, i furbetti. Il beneficio è condizionato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, i quali dovranno sottoscrivere il patto per il lavoro presso i centri per l'impiego e rispettarne gli obblighi. Per questo abbiamo previsto il potenziamento dei centri per l'impiego che, nell'indifferenza generale di tutti i Governi passati (nessuno escluso), operano in condizioni difficili e, anzi, impossibili da decenni. I dati Eurostat sulla spesa per i servizi pubblici per l'impiego evidenziano un disarmante divario rispetto agli altri Paesi europei: nel 2015 L'Italia ha speso un terzo della Spagna e un sesto rispetto alla Francia. Per la prima Per la prima volta un Governo investe seriamente sul sistema delle politiche attive impegnando ben 2 miliardi di euro nel prossimo biennio. Signor Presidente, Basta con l'austerità che abbatte crescita e diritti. Adesso pensiamo ai più deboli; mettiamo al primo posto il diritto al reinserimento, la dignità, il lavoro e i lavoratori; investiamo sulla produttività del Paese, scommettendo sulla formazione di milioni di persone e sulla valorizzazione del capitale umano. Come siamo arrivati a fare tutto questo? Abbiamo semplicemente tratto insegnamento dal passato e dalla triste esperienza maturata, subendo il malgoverno degli anni scorsi. Quei Governi, con questo provvedimento sul reddito di cittadinanza e quota 100, saranno condannati all'oblio perché un buon legislatore trae sempre insegnamento dai risultati nefasti dei Governi passati per non fare gli stessi errori. La storia insegna - come disse e scrisse una volta il grande scrittore Günter Grass - ma per trarne gli insegnamenti giusti bisogna essere dei buoni allievi.

abbia l'opposizione contro i poveri. Negli interventi dei colleghi della minoranza oggi ho registrato scenari nefasti e velleità vaticinanti degni dell'oracolo di Delfi che prefigurano crisi a causa di un provvedimento ancora in discussione e non ancora approvato. Io non lo capisco. I colleghi dell'opposizione dispensano consigli; lo hanno fatto anche in Commissione. Offrono a noi ricette per migliorare il provvedimento. Con queste ricette, però, hanno cucinato e - direi - bruciato le pietanze e le speranze di milioni di italiani quando erano loro al Governo.

da una parte abbiamo i sostenitori del reddito di cittadinanza che si guardano bene dal parlare e dal sostenere quota 100, e dall'altra abbiamo i sostenitori di quota 100 che si guardano bene dal sostenere il reddito cittadinanza.

Il reddito cittadinanza è un sussidio vero e proprio, è una forma di assistenzialismo fine a sé stessa, tanto che affidate ai centri per l'impiego

colleghe e colleghi, oggi è un giorno grandioso non solo per attivisti, simpatizzanti e portavoce del MoVimento 5 Stelle, ma per tutta l'Italia. Infatti siamo in quest'Aula per approvare finalmente un provvedimento che mette al centro i bisogni, i diritti e la dignità dei cittadini italiani. Fin dal suo primo ingresso in Parlamento, sei anni fa, il MoVimento si è battuto per l'istituzione del reddito di cittadinanza. Abbiamo fatto marce e manifestazioni, ed ora sta per diventare realtà. Da mesi ci sentiamo dire che il reddito di cittadinanza è una misura assistenzialista e favorirà coloro che non vogliono lavorare: niente di più sbagliato. Gli italiani non sono come li dipingete, fannulloni pronti a tutto pur di stare a casa seduti sul divano.

I nostri concittadini che negli ultimi anni hanno perso il lavoro sono disperati: imprenditori e padri si sono suicidati perché non sapevano come andare avanti. Con il reddito di cittadinanza offriamo un'ancora di salvezza, nell'attesa di trovare un nuovo lavoro, a chi non chiede altro che riconquistare la dignità alzandosi al mattino per andare a lavorare e vivere del proprio lavoro. Ma parliamo dei numeri di questo provvedimento, visto che tante polemiche sono sorte intorno a questi. Si dice che sia una misura fatta a beneficio del Sud, ma in realtà il 47 per cento dei beneficiari vive al Centro-Nord. Il reddito è atteso da tutti, da Nord a Sud. Parlo ad esempio della mia Regione, il Piemonte, che ha subito molto più di altre aree del Nord la crisi degli anni passati; i tassi di disoccupazione sono ancora oggi per circa un terzo superiori rispetto a queste. Chi crede che al Nord il reddito vedrà poche richieste si sbaglia o vive in un altro mondo. Ovunque c'è bisogno di un sostegno che aiuti chi si è trovato in difficoltà, di centri per l'impiego efficienti e di figure in grado di aiutare nel percorso di riqualificazione. Per questo l'introduzione del reddito di cittadinanza è accompagnata dalla riforma delle politiche attive del lavoro che passa anche per l'assunzione di 10.000 nuove unità di personale presso i servizi per l'impiego. Finalmente l'Italia si dota di uno strumento di *welfare* presente da tempo in quasi tutti i Paesi dell'Unione europea. E non credete a chi vi racconta che era già stato fatto con l'introduzione del Rei, visto che questa misura era rivolta a una platea estremamente ridotta rispetto ai 5 milioni di poveri

che invece consentirà ai percettori di uscire dalla soglia di povertà assoluta e ricominciare a condurre una vita dignitosa. Ma in questo provvedimento non c'è solo il reddito, ci sono anche le misure di uscita anticipata dal lavoro, per poter finalmente rompere le inique catene imposte dalla legge Fornero. E mi riferisco a quota 100 (già ampiamente descritta dai colleghi) ma ancor più ad opzione donna. Negli ultimi mesi siamo stati tutti bersaglio di campagne sui *social* per portare alla nostra attenzione la richiesta di prorogare questa misura che tanto aveva trovato il favore delle donne, che hanno così la possibilità di andare in pensione

Alcune colleghe ed io abbiamo depositato un ordine del giorno che impegna il Governo a reperire le risorse per estendere la misura anche per gli anni a venire, così da dare la possibilità di ritirarsi dal lavoro anche a quelle donne rimaste fuori dal provvedimento per una manciata di mesi. Quindi - e concludo - con le misure contenute in questo decreto andiamo a porre un altro fondamentale tassello nella trasformazione del nostro Paese, dopo il decreto dignità - che, per inciso, si sta rivelando straordinariamente efficace nel promuovere la stabilizzazione

Finalmente offriamo a tante persone - come ad esempio alla signora Rosa, che tante volte preoccupata in questi mesi mi ha scritto e persino telefonato - la possibilità di andare in pensione prima, per potersi godere i nipoti. Offriamo ai nostri giovani la possibilità di entrare fattivamente nel mondo del lavoro, ma soprattutto consentiamo a milioni di cittadini di rialzare la testa e di rimettersi in gioco. Ci sono voluti anni di battaglie, dentro e fuori dai Palazzi, ma alla fine, come si dice, chi la dura la vince. E a vincere oggi sono i cittadini.

in premessa la difficoltà di fare questo intervento, perché non vorrei essere nei panni delle opposizioni, in modo particolare del PD, ma anche degli amici di Forza Italia, e quindi non vorrei condividere la loro frustrazione politica nel vedere demolito, con questo provvedimento, ciò che loro hanno approvato insieme, cioè la legge Fornero *(Applausi avrebbero voluto fare (Forza Italia) e che hanno fatto senza grandi successi in merito al reddito di cittadinanza. In tanti ci dicevano che non si può fare. Come contraltare allo *slogan* della Lega «stop Fornero», in tanti dicevano che non si può fare. E noi lo abbiamo fatto. Oggi questa maggioranza fa ciò che in tanti volevano scoraggiarci dal fare, perché bisognava salvaguardare, a spese dei cittadini, le patrie casse. Si può fare e anzi si deve fare questo provvedimento, perché la legge Fornero è un provvedimento che è stato approvato contro il popolo e ogni provvedimento che viene approvato contro il popolo deve essere bocciato. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. È contro il popolo un provvedimento che aumenta inopinatamente l'età pensionabile ed è contro il popolo un provvedimento che, per esempio, crea quella sacca di diseredati che sono appunto gli esodati, i figli di nessuno; è contro il popolo un provvedimento che punta a mortificare le persone e i cittadini. La bontà di questa nostra scelta è dovuta al fatto che siamo consapevoli questo è l'inizio di un percorso. Come dice sempre Salvini, noi stiamo demolendo la legge Fornero; l'obiettivo è quello di arrivare, da qui a tre anni, a quota 41. 41. La bontà di questo percorso è testimoniata in maniera oggettiva e indiscutibile non dalle chiacchiere del politichese, ma dalla formidabile adesione che tantissimi cittadini, migliaia e migliaia di cittadini italiani, hanno manifestato nei confronti di quota 100. È un percorso importante, che fa il paio con il reddito cittadinanza. Il collega Tosato prima l'ha detto: noi abbiamo un paradosso in questa Aula, dove le opposizioni legittimamente avversano il reddito di cittadinanza. Da una parte abbiamo il PD e il centrosinistra, che lo fanno dopo aver fallito con il reddito di inclusione, e dall'altra gli amici di Forza Italia, che lo fanno dopo che in campagna elettorale hanno sbandierato a più non posso il reddito di dignità. Noi invece facciamo quello che abbiamo promesso, e lo facciamo non per fare accomodare gli italiani. Chi dice che questa misura, così come è arrivata in Parlamento, tende a favorire l'assistenzialismo dice qualcosa che non corrisponde al vero. Il reddito di cittadinanza uscirà da questo Parlamento, dal Senato e dalla Camera, in in maniera strutturata e collegata con un percorso lavorativo, perché noi vogliamo dare una prospettiva agli italiani e non vogliamo assolutamente fare in modo che gli italiani possano perdere fiducia verso lo Stato e verso il loro Paese.

e radicalmente diverso rispetto a quelli seguiti da coloro che hanno governato il Paese fino a qualche mese fa perché noi proviamo a dare all'Italia e agli italiani una nuova vita, agli anziani una nuova vita che va lungo il percorso della dignità perché chi ha lavorato per una vita intera, chi si è spaccato la schiena per una vita intera, chi ha condotto la propria vita personale e familiare a testa alta, faticando per portare a casa uno stipendio, è giusto che ad una certa età possa godersi la famiglia, la moglie, i nipoti

che si chiama speranza perché quota 100, e anche il reddito di cittadinanza, al di là delle congetture strumentali e politiche, tendono a dare nuove opportunità di lavoro perché se in tanti andranno in pensione, in tanti avranno una nuova *chance* e in tanti ritorneranno a vivere. È un dato oggettivo inequivocabile che non si può smentire. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Per concludere, a queste persone, agli anziani che potranno godersi la loro vita con dignità e ai giovani che potranno percorrerla, invece, con speranza, dobbiamo anche dedicare un pensiero e cioè che quelle lacrime

questo intervento con un caloroso saluto: *bye bye* Fornero, senza rancore, ma senza rammarico.

Signor Presidente, non avrei mai pensato che il 2019 potesse diventare un anno storico - forse ancor più del 2018 del 2018 - perché finalmente si è posata una pietra miliare contro la povertà, una piaga che affligge e che ha afflitto molte famiglie italiane in qualsiasi epoca della nostra storia. L'approvazione del decreto sul reddito di cittadinanza, e principalmente la sua conversione in legge che spero arriverà tra pochi giorni in queste Aule, è e rappresenta un atto concreto contro la povertà, contro le diseguaglianze, contro l'umiliazione che ha subito e subisce chi purtroppo non ha le risorse necessarie per vivere e ora ha a disposizione la possibilità di ripartire. Un atto di coraggio, certo, di grandioso coraggio hanno avuto i nostri colleghi di Governo che hanno approvato in modo ampiamente condiviso questo decreto. Eravamo gli ultimi nel campo degli strumenti contro la povertà. Dappertutto hanno misure simili al reddito di cittadinanza, in linea con il comma 3 dell'articolo 34 della Carta europea dei diritti fondamentali. Ma su questo l'Europa non vigila come su altri aspetti. Difatti, questa Unione della quale facciamo parte, basata sui trattati, sugli accordi internazionali, sui paletti da rispettare, sulle soglie da non superare, sulle direttive da recepire, sulla concorrenza, sul commercio, sul mercato, sulle banche, su tutte queste cose per le quali siamo sorvegliati speciali e non possiamo sbagliare e per le quali rischiamo ogni giorno di andare incontro a sanzioni pesanti per le casse dello Stato e per i cittadini, questa Europa, alla voce povertà, che è persino riconosciuta nella Carta fondamentale dei diritti dell'uomo

Presidente, si tratta di scelte. I Governi precedenti hanno scelto di liberalizzare in modo selvaggio il mercato del lavoro con lavori più facili da dare, più difficili da tenere, con meno diritti e più doveri, con più facilità di entrare e uscire, di assumere, di licenziare, lavoro a chiamata, lavoro facile, forse per i datori ma non per i lavoratori. Un lavoro così precario da essere inconciliabile con una vita serena, con uno stipendio costante, con un'entrata certa, con la possibilità di programmare e di fare progetti, di mettere su famiglia, di fare figli, di acquistare una casa. una liberalizzazione del mercato del lavoro che ha incrementato la povertà. Colleghe e colleghi, queste affermazioni sono basate su studi che dimostrano come vi sia una relazione diretta tra la liberalizzazione del mercato del lavoro e la povertà. Lo dimostrano i dati, i numeri, i grafici. Lo dimostrano i fatti. Tanto che in un nucleo familiare lo stato di povertà peggiora in modo più marcato con la presenza di un lavoratore precario rispetto alla presenza di una persona disoccupata. In altre parole, pesa di più l'incertezza di una paga inferiore alle aspettative e discontinua rispetto alla possibilità del disoccupato di trovare un lavoro stabile. Ebbene, Presidente, gli Stati sul problema della povertà sono liberi di fare scelte e in Italia ci siamo forse distratti un po' troppo, abbiamo forse aspettato un po' troppo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. In dieci anni i poveri assoluti sono passati da un milione a 5 milioni. La povertà è un problema serio. Probabilmente il problema più serio per un Paese avanzato. Un problema che, a mio modestissimo giudizio, presenta due sfaccettature; una prettamente economica e una riferita alla miriade di criticità che spesso incontrano le persone che si trovano in quello stato. Per la parte economica vi è senza dubbio l'assenza di un'occupazione, di un lavoro stabile e regolare, di uno stipendio adeguato per permettere una vita dignitosa. Sicuramente, in parte, questo è dovuto al fatto che le possibilità occupazionali spesso sono inferiori alle richieste, alle aspettative, soprattutto nelle zone poco fertili dal punto di vista imprenditoriale e per gli investimenti. Se vi è poco lavoro, sono poche le persone che hanno competenze sufficienti per potersi accaparrare quel posto di lavoro. Colleghi, colleghe, Presidente, è però solo un problema di competenze, capacità e preparazione? La risposta è no, perché molte persone che versano in stato di povertà hanno anche altri tipi di problemi di natura sociale, familiare, culturale, oltre a criticità che hanno a che fare con la salute, l'abitazione, la chiusura in se stessi, l'assenza di voglia di vivere e l'impossibilità di affrontare i problemi quotidiani. Una molteplicità di problemi così vasta da rendere difficile trovare soluzioni adeguate per le quali serve un'assistenza e un'analisi differenziata, completa e integrale. Per tale ragione il reddito di cittadinanza prevede diversi approcci a seconda delle criticità della persona; da una parte il percorso prettamente occupazionale per chi non ha difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro e, dall'altra, percorsi di inclusione sociale finalizzati ad alleviare le sofferenze di chi va aiutato. Non dobbiamo pensare che sia tutto così facile, ma prima o poi la macchina andava messa in moto, *in primis* per le persone che avevano bisogno di un maggiore impegno da parte delle istituzioni. Il reddito di cittadinanza è una misura valida e concreta contro la povertà perché comprende soluzioni diverse per problemi diversi: il sostegno economico è forse la cosa più importante, ma non sufficiente per uscire dal disagio. Per questo si è puntato molto sul lavoro e sui percorsi formativi e occupazionali, così come si è puntato molto sugli incentivi che in modo completo e differenziato faciliteranno l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e per migliorare il più possibile l'aspetto formativo. Sono infatti previsti incentivi per le aziende che assumono, per i *tutor* e le agenzie pubbliche e private che collocano il beneficiario, per le agenzie di formazione che fanno e faranno corsi utili, una volta per tutte. E, ancora, per i beneficiari che avviano un'attività imprenditoriale in modo autonomo sono previsti incentivi premianti e, forse, questa è veramente la cosa più importante. Il reddito di cittadinanza fa bene a chi sta peggio e fa bene anche alla nostra economia; è la pietra angolare da cui l'Italia può ripartire. Oggi con il reddito di cittadinanza possiamo considerarci al pari dei nostri *partner* europei e faremo vedere che anche l'Italia è pronta per un cambiamento culturale fatto di sensibilità, di solidità di altruismo e pragmatismo, di serenità e di lavoro, di contributi, di controlli, di gentilezza e severità, di maniche arrotolate e di abbracci tra persone che hanno scelto una volta per tutte di voler bene, più bene a chi per troppo tempo è rimasto indietro. *(Applausi

che il problema fondamentale del nostro tempo sia la disuguaglianza è certamente un elemento chiaro e che questa disuguaglianza sia anche segno e responsabilità della globalizzazione per come è avvenuta, del fallimento delle politiche di austerità europea e in questo anche delle responsabilità che il centrosinistra in Europa ha avuto in questi anni, è un dato acquisito.

e chiaramente non condivido l'idea secondo la quale se si fa un intervento sulla povertà lo si fa per i fannulloni che stanno sul divano. Sono affermazioni che non condivido e che considero profondamente sbagliate. Detto questo, questo, faccio un'altra precisazione, perché è troppo semplice il confronto tra propaganda e parole: non condivido nemmeno l'obiezione secondo la quale un reddito di 780 euro produrrebbe un problema per chi ha un lavoro e ha salari più bassi.

lotta alla povertà - che, ripeto, è giusta - e politiche attive per il lavoro. È una cosa che purtroppo non funzionerà, per alcune ragioni statistiche.

non avrà la possibilità del lavoro, non perché non lo trova, ma perché non può andare a lavorare. Come affrontiamo, dunque, tale questione?

con le politiche sociali gestite in primo luogo dai Comuni, e dall'altra le politiche attive per il lavoro.

il fatto che siete in una situazione di conflitto con le Regioni e con gli enti locali, su cui scaricate una serie di competenze e che non avranno né le risorse,

Possibile che in questo dibattito non vi sia nessuna relazione reale tra le politiche di sostegno e le politiche di inserimento lavorativo? Qui il problema è che non si produce lavoro e che ci troviamo all'interno di un processo recessivo. Sono colpito dal fatto che nessuno di voi abbia nemmeno dialettizzato questo problema.

andando? Voi parlate di diritti, avete citato Gramsci - e lo apprezzo - avete parlato del bene comune, avete messo davanti i più deboli,

porterà una parte di queste famiglie a non poter accedere al reddito perché non potranno avere i documenti che state chiedendo, e lo sapete. Per non parlare delle persone senza fissa fissa dimora e dei minori. Insomma, c'è una serie di problemi che questo provvedimento non è in grado di risolvere.

patteggiamento, a tappare le orecchie rispetto al dibattito e a cercare la mediazione tra di voi. Ma questo non sarà quel miracolo che voi avete annunciato qui per il nostro Paese.

Signor Presidente, prima di entrare nel vivo del mio intervento vorrei ricordare a tutti coloro che oggi siedono in quest'Aula e che a suo tempo hanno votato a favore della legge Fornero che noi della Lega quella schifezza non l'avevamo votata. Riguardo ad alcuni interventi, che ho seguito con attenzione, di colleghi delle opposizioni, di colleghi delle opposizioni, che sembrano al ballo delle debuttanti, dimenticandosi dei danni che hanno fatto, dal mio punto di vista sarebbe stato più appropriato un doveroso silenzio. però, che sono voluto intervenire, mi permetto di sottolineare che, se avessi avuto l'occasione di dar loro un consiglio avrei suggerito dei semplici concetti di base. Prima di iniziare gli interventi, avrei suggerito loro di guardare per una volta fisso nella telecamera, senza ricorrere ai soliti lunghi *show* mediatici per guadagnare un po' di attenzione, avrei suggerito loro di fare un respiro e, per una volta, rivolgersi a tutti i giovani a cui hanno rubato il futuro, a tutti gli esodati e alla gente che è stata rovinata dalla loro sciagurata legge. A questo punto, se avessero voluto dire qualcosa di veramente intelligente agli italiani, sarebbero bastate tre semplici e umili paroline, che nelle Aule dei palazzi si sentono veramente poco: «Scusateci, abbiamo sbagliato». Io non ho dimenticato, nessuno di noi qui ha dimenticato e nemmeno il popolo italiano fuori da quest'Aula ha dimenticato e mai dimenticherà: 6 dicembre 2011, conversione in legge del decreto-legge n. 201, articolo 24, la data infelice che passerà alla storia come il giorno in cui il Governo Monti e la maggioranza che allora lo sosteneva hanno ferito il popolo italiano in maniera quasi mortale, con un provvedimento vigliacco profondamente ingiusto quale la riforma Fornero. *(Applausi Mi ricordo bene quel periodo in cui c'era il Governo dei tecnici: quelli bravi, che piacevano tanto all'Europa e che dicevano di voler salvare l'Italia, che oggi non sono neanche qua seduti, ma magari sono a casa a guardarci quelli che dicevano di salvare l'Italia, ma che in realtà stavano facendo l'esatto contrario. *(Applausi quando ero io a stare casa a sentire l'allora ministro Fornero pronunciare la fastidiosa parola *choosy*, per definire i giovani italiani come me.

una generazione che sta facendo ogni tipo di lavoro per sopravvivere, questa: una generazione di diplomati e laureati con più *master* che soldi in tasca, di persone ritenute troppo vecchie per lavorare per più di tre anni nello stesso posto con stipendi da fame e nessuna tutela e, al contempo, ritenute troppo giovani, perché oggi se ne cercano con esperienza anche per cucinare i panini in un *fast food* o in un bar. *(Applausi dai

Meno male che sono arrivati la Lega di Salvini e questo Governo! Per fortuna, oggi finalmente riusciamo a voltare quella brutta pagina di politica del nostro Paese. Per fortuna, oggi finalmente possiamo ridare ai lavoratori e alle prossime generazioni di lavoratori la speranza di andare in pensione ad un'età consona, per potersi godere la propria vecchiaia. Per fortuna, oggi finalmente ridiamo dignità ai lavoratori precoci, a coloro che fanno lavori usuranti, alle donne e ai più deboli. D'ora in poi andare in pensione diventerà una scelta, non più la rincorsa di una meta sempre più distante. Grazie a Matteo Salvini, alla Lega e a questa maggioranza di Governo, 100 non è più una promessa, ma da oggi è una realtà, una scelta: la libera scelta di andare in pensione dopo una vita passata a lavorare.

Si può fare di meglio? Certo, si può sempre fare di meglio e siamo sempre a disposizione dei cittadini per fare di meglio, ascoltare le loro esigenze e risolvere i loro problemi. Questo per noi è fare politica. Con il nostro sistema pensionistico, la pensione non sarà cumulabile con altri redditi da lavoro, perché vogliamo favorire quel ricambio generazionale che ci avete negato. Vogliamo dare ai giovani l'opportunità di entrare nel mondo del lavoro, guadagnare, fare una famiglia, progettare il proprio futuro con maggior serenità e senza la paura del domani. Abbiamo inserito l'opzione donna per le lavoratrici dipendenti a cinquantotto anni e a cinquantanove per le autonome con almeno trentacinque anni di contributi. Abbiamo applicato ai lavoratori precoci gli adeguamenti sulla speranza di vita; abbiamo inserito il TFS per tutti i pensionati pubblici e non solo per quelli di quota 100, quindi si ha la possibilità di avere subito l'anticipo del TFR fino a 45.000 euro, Questo è un cambio di rotta: con quota 100, i latitanti finalmente vedranno sospesa la loro pensione; anche per loro sono finiti i tempi della pacchia. Siamo orgogliosi di questo provvedimento, che è una risposta concreta agli italiani: questo ci chiedeva la gente, niente più *choosy*, niente più lacrime, niente più riforme che piacciono più ai burocrati europei che ai lavoratori italiani. Non un regalo o uno *spot* elettorale, ma una legge giusta per andare in pensione. Ancora una volta, la Lega di Matteo Salvini e questo Governo passano dalle parole ai fatti, ecco il vero cambiamento: questo significa avere contatto con la realtà e con il Paese, mentre c'erano Governi che mettevano come priorità le banche, le cooperative, le *lobby*, lo *ius soli*, le adozioni *gay*, il genitore 1 e il genitore 2. Noi no. Noi ci occupiamo della vita quotidiana delle persone, dei problemi reali. Il resto lo lasciamo agli altri o a quel che resta degli altri. A dir la verità, questa sera è rimasto ben poco degli altri, però fa nulla. Il vostro essere continuamente slegati dalla realtà, definendoci con disprezzo populisti e sovranisti, per me è soltanto una medaglia sul petto che metterò vicino alla legge sulla legittima difesa e al decreto-legge sicurezza e, da oggi, a quota 100. Perché, da quando siete all'opposizione, avete finito di fare danni e avete finito di rubarci il futuro.

Lo fa con quasi trent'anni di ritardo e lo fa grazie al lavoro e all'ostinazione del MoVimento 5 Stelle. nel 1992 l'Europa chiese all'Italia di introdurre delle misure sul reddito garantito. Più precisamente, la raccomandazione del Consiglio 92/441, in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale recita al dodicesimo punto: «(...) il Parlamento europeo, nella sua risoluzione concernente la lotta contro la povertà nella Comunità europea, ha auspicato l'introduzione in tutti gli Stati membri di un reddito minimo garantito, inteso quale fattore d'inserimento nella società dei cittadini più poveri». *(Applausi dal Gruppo M5S)*. L'accesso al reddito minimo garantito, secondo le raccomandazioni dell'Unione europea, dovrebbe essere rinnovabile, senza restrizioni temporali. Tale diritto avrebbe un carattere ausiliario rispetto agli altri diritti sociali e alle altre politiche, per favorire l'integrazione economica e sociale. Perché dico questo? Perché mentre venivo qui questa mattina, ho ripensato a tutto quello che è successo in questi anni. È successo tanto, è successo di tutto. È successo che un movimento di cittadini, nato e cresciuto senza soldi pubblici, nelle piazze, tra la gente è arrivato in meno di dieci anni al Governo del Paese. E una volta lì, ha rispettato gli impegni presi con i cittadini. Per qualcuno questa è una cosa strana, infatti si cerca sempre il modo di sminuire quello che di buono stiamo facendo. Invece per noi si chiama e si chiamerà sempre coerenza. Qualcuno in quest'Aula ha detto che con questo provvedimento noi stiamo finanziando il nulla. Il nulla? Restituire dignità a cinque milioni di persone che, a causa della crisi, sono rimaste indietro e che sono in povertà assoluta è il nulla? Non fateci ridere, per favore. Con il reddito di cittadinanza non facciamo altro che dare attuazione ai principi sanciti dalla Costituzione, a lungo rimasti inapplicati, e alle raccomandazioni dell'Unione europea. E lo facciamo mettendo al centro l'occupazione: l'investimento in politiche attive per il reinserimento nel mondo del lavoro, attraverso la riorganizzazione dei centri per l'impiego, è uno degli elementi qualificanti di questa misura. Dal PD obiettano che il reddito di cittadinanza è una fotocopia del Rei, ma non c'è niente di più sbagliato. Il precedente Governo ha trascurato gli investimenti in politiche attive, in formazione e in personale che seguisse il disoccupato per il reinserimento nel mondo del lavoro. Con il reddito di cittadinanza, al contrario, il sostegno al reddito è strettamente legato al percorso formativo attraverso i centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro, gli enti di formazione, i servizi sociali dei Comuni e le Regioni. Dal 2013, da quando abbiamo depositato il primo disegno di legge sul reddito di cittadinanza a prima firma dell'ostinatissima presidente della Commissione lavoro Nunzia Catalfo, non ci siamo fermati un giorno. *(Applausi Abbiamo dato battaglia nelle Aule parlamentari e nelle Commissioni. Abbiamo fatto i banchetti nelle piazze. Abbiamo marciato insieme a migliaia di persone che arrivavano da tutta Italia: una marea umana di uomini uomini e donne che in questi anni ci ha sempre fatto sentire il proprio, fondamentale sostegno. Ecco, le donne. Lo voglio dire oggi, davanti a tutti voi: il reddito di cittadinanza è una misura che pone un'attenzione altissima sulle donne. A maggior ragione, visto che l'Italia - e questo non lo dico io, ma lo dice un rapporto del World economic forum sul Global gender gap - è il Paese con il più alto numero di donne iscritte all'università, ma, allo stesso tempo, fanalino di coda per occupazione femminile. Proprio così: un circolo vizioso che dobbiamo assolutamente spezzare e per farlo il reddito di cittadinanza è un elemento importantissimo. Infatti - lo ricordo a chi evidentemente non ha studiato il provvedimento ma si ostina a volerci dare lezioni, malgrado i suoi memorabili fallimenti - questa è una misura per il lavoro, una misura per il lavoro, equa, giusta, di vera emancipazione, visto che alle donne viene riconosciuto un ruolo assolutamente paritario all'interno del nucleo familiare, che percepisce il reddito di cittadinanza attraverso il meccanismo della quota parte. Sarà un'occasione di vero riscatto per quelle tantissime donne che abbiamo incontrato in questi anni e che ci hanno raccontato le loro difficoltà, le paure, i progetti che avrebbero voluto realizzare per loro e per i loro cari, ma che si sono infranti contro le difficoltà che comporta il non avere un impiego. Adesso queste donne vedranno lo Stato schierarsi veramente dalla loro parte, tendendo loro la mano e accompagnandole in un serio e costante percorso di formazione e riqualificazione. Ma non solo; perché, come previsto dal decreto-legge, a coloro che vorranno intraprendere un lavoro autonomo, avviare un'impresa individuale o una società cooperativa nel primo anno di erogazione del beneficio saranno riconosciute sei mensilità di reddito di cittadinanza, che saranno versate in un'unica soluzione. Allo stesso tempo, però, abbiamo voluto riconoscere i compiti di cura delle madri con figli di età inferiore ai tre anni, che saranno escluse dal percorso di condizionalità previsto per chi beneficia del reddito di cittadinanza. Si è intervenuti, infine, sulle famiglie con disabili, che rientravano nella platea dei beneficiari già nella stesura originaria del decreto-legge. La tutela è stata ulteriormente rafforzata: per esempio, il familiare di un disabile grave o non autosufficiente sarà esonerato dagli obblighi previsti per ottenere il reddito ma, se vorrà aderire al patto per il lavoro, potrà comunque farlo. Un atto dovuto, in attesa di approvare altri importanti provvedimenti, come quello per il riconoscimento e il sostegno del *caregiver* familiare, già calendarizzato in Commissione Commissione lavoro (è già partito). Perché questo - lo ribadiamo e lo ribadiremo sempre - è un Governo di cittadini per i cittadini.